L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sulle ulteriori iniziative in relazione all'emergenza da Covid-19». Ha facoltà di parlare il presidente del Consiglio dei ministri, professor Conte. Gentile Presidente, onorevoli senatrici e onorevoli senatori, riferisco oggi in Senato in vista dell'imminente scadenza dello stato d'emergenza che, in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, fu deliberato in Consiglio dei ministri il 31 gennaio per la durata di sei mesi (quindi viene a scadere alla fine di questo mese). Pur in assenza di un vincolo normativo, ritengo doveroso condividere con il Parlamento questa decisione. Si è concluso poche ore fa

Ricordo che la dichiarazione dello stato d'emergenza è prevista dal codice della Protezione civile (che è una fonte di rango primario di carattere generale

per l'attivazione di una serie di poteri e facoltà necessari per affrontare con efficacia e tempestività le situazioni emergenziali in atto.

Quel potere d'ordinanza consente infatti di emanare norme in deroga a ogni disposizione vigente, ovviamente nei limiti con le modalità indicati nella deliberazione dello stato d'emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico delle norme dell'Unione europea. La decisione che l'Esecutivo intende assumere trova quindi la sua fonte di legittimazione nell'articolo 24 del decreto legislativo n. 1 del 2018, che, sempre con delibera del Consiglio dei ministri, consente la proroga dello stato d'emergenza fino a una durata massima di dodici mesi.

Quest'esigenza - e qui faccio una notazione statistica - si verifica quasi sempre, come confermano molteplici precedenti: lo stato d'emergenza viene ordinariamente prorogato dal Governo ben oltre il termine inizialmente fissato. Segnalo, ad esempio, che dal 2014 ad oggi sono state adottate 154 dichiarazioni di stato di emergenza e ben 84 sono state le delibere di proroga. Sarebbe, d'altra parte, incongruo - se ci pensate - sospendere bruscamente l'efficacia delle misure adottate, se non quando si siano compiutamente esauriti i procedimenti avviati e la situazione, in base a criteri di ragionevolezza e proporzionalità, sia riconducibile a un tollerabile grado di normalità. Se questo è vero per eventi che si esauriscono una volta per tutte (pensate a un terremoto, a un'alluvione), lo è ancor di più in questo caso, per un evento come la pandemia che non si è risolto in un fatto puntuale, ha assunto i tratti di un processo in continua, imprevedibile evoluzione e che purtroppo ancora oggi, seppure in misura contenuta, territorialmente circoscritta, non ha completamente esaurito i suoi effetti. Se decidessimo diversamente, se ci assumessimo la responsabilità di non prorogare lo stato di emergenza dichiarato il 31 gennaio scorso, dobbiamo essere consapevoli

A puro titolo di esempio cito alcune delle misure che perderebbero *ex abrupto* la loro efficacia: l'allestimento e la gestione delle strutture temporanee per l'assistenza alle persone risultate positive; l'impiego del volontariato di Protezione civile; il reclutamento e la gestione di *task force* di personale sanitario a supporto delle strutture regionali e - attenzione - degli istituti penitenziari; la prosecuzione dell'attività relativa al numero verde 1500 per l'assistenza alla popolazione; il pagamento dilazionato delle pensioni presso gli uffici postali per evitare assembramenti; l'attribuzione all'Istituto superiore di sanità della sorveglianza epidemiologica. Menziono inoltre l'attivazione del sistema CROSS, di cui forse non riconosciamo comunemente l'importanza. CROSS sta per Centrale remota operazioni di soccorso sanitario: in caso di mancanza di posti letto nei reparti di terapia intensiva di una Regione, quando c'è sovraffollamento, CROSS interviene per prevedere - dopo il nostro intervento normativo, addirittura obbligatoriamente - la ripartizione e il trasferimento dei pazienti in ospedali situati in altre Regioni. Tra le misure che perderebbero efficacia vi è anche quella che consente di noleggiare navi per la sorveglianza sanitaria dei migranti e non sfugge a nessuno quanto sia attuale quanto sia attuale il ricorso a questo strumento che concorre, insieme agli altri apprestati dalle autorità, a un ordinato svolgimento della quarantena a tutela della sanità pubblica. Proprio a tale riguardo, infatti, gli uffici e le strutture dei Ministeri competenti sono intensamente impegnati a far fronte a una situazione complessa, che va affrontata con risoluzione, efficacia e tempestività. Siamo veramente convinti di voler interrompere tutte queste attività? Ne ho citate alcune a titolo esemplificativo. Non solo, se lo stato di emergenza non fosse prorogato, cesserebbe la funzione di coordinamento attribuita al capo della Protezione civile, così come decadrebbero i poteri straordinari attribuiti ai molteplici soggetti attuatori, designati per l'espletamento di una miriade di specifici compiti, che non vi sto ad elencare. I soggetti attuatori per la maggior parte dei casi sono i Presidenti delle Regioni, oltre che il Segretario generale del Ministero della salute e i soggetti attuatori responsabili della gestione della sorveglianza sanitaria dei migranti. Verrebbe a cessare le proprie funzioni anche il comitato tecnico-scientifico, che in questi mesi - è noto a tutti - ha svolto un ruolo importante nel sostenere e motivare con evidenze scientifiche scientifiche le decisioni del Governo, sia nella fase della progressiva limitazione delle relazioni di comunità e della sospensione delle attività economiche e commerciali, sia nella delicata fase della loro graduale riapertura e del progressivo ritorno alla normalità. A questo occorre poi aggiungere che al 31 luglio, data di cessazione dello stato di emergenza, sono correlati numerosi termini contenuti in provvedimenti normativi di rango primario, e anche secondario, adottati durante lo stato di emergenza. Com'è noto, molte disposizioni assumono come riferimento temporale della loro efficacia la cessazione dello stato di emergenza - si tratta, quindi, di un riferimento temporale *per relationem* - mentre altre prevedono termini di efficacia a date diverse, ma comunque anche in questo caso determinate *per relationem* alla data di scadenza dello stato emergenziale. Anche qui faccio un esempio per essere ancora più chiaro e cito per tutte una disposizione emblematica, l'articolo 122

Quindi, la mancata proroga dello stato di emergenza finirebbe per far cessare l'operatività del commissario, il cui lavoro, accanto a quello della Protezione civile, si sta rivelando fondamentale. La struttura commissariale, infatti, sta continuando a svolgere i suoi compiti, con particolare riguardo alla produzione e alla distribuzione di beni strumentali utili a contenere e a contrastare l'emergenza - parliamo ovviamente delle note apparecchiature e dei dispositivi medici di protezione individuale - ma anche al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere, con specifico riferimento ai reparti di terapia intensiva e subintensiva, nonché al rafforzamento delle filiere produttive dei beni necessari per il contrasto all'emergenza. Sta inoltre ponendo in essere un'importante attività di sostegno al Ministero della giustizia per assicurare il regolare svolgimento delle attività processuali, rese difficili, com'è noto, com'è noto, dalle esigenze di distanziamento. Soprattutto in questa fase la struttura commissariale sta procedendo all'acquisizione e alla distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, nonché di ogni altro bene strumentale, compresi gli arredi utili a garantire per settembre utili a garantire per settembre l'ordinato avvio dell'anno scolastico. *(Commenti).* Sono più di 10 milioni le persone, tra studenti, insegnanti e personale amministrativo, che dovranno rientrare nelle scuole nella massima sicurezza ed è obiettivo da tutti riconosciuto come prioritario. Ovviamente le forze di maggioranza e di opposizione si uniscono verso questo obiettivo obiettivo che, per essere raggiunto, richiede uno sforzo molto elevato, uno sforzo anche collettivo in termini di organizzazione, di rapido reperimento di spazi e strumentazioni adeguate. È una grande sfida per il Paese. Parimenti correlate alla data del 31 luglio sono anche le misure previste dal decreto-legge n. 33 del 2020, il cosiddetto decreto-legge riaperture. Ai sensi dell'articolo 3 di tale decreto, le misure si applicano, salvo eccezioni, dal 18 maggio al 31 luglio 2020. Tra le misure in questione figurano anche specifiche prescrizioni comportamentali che sono risultate e risultano decisive per il contenimento del contagio: ad esempio, il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, l'obbligo di assicurare il mantenimento della distanza di almeno un metro nelle riunioni. Benché la proroga dello stato di emergenza non sia - questo bisogna dirlo anche molto chiaramente - condizione di legittimità per estendere temporalmente l'efficacia delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza, è tuttavia evidente che, in concreto, i presupposti di carattere sostanziale che giustificano la proroga delle disposizioni contenute nei decreti-legge nn. 19 e 33 del 2020, si radicano, come ritiene la migliore dottrina costituzionalistica, proprio nella dichiarazione dello stato di emergenza. Rinnovare quelle misure, infatti, senza prorogare lo stato di emergenza, esporrebbe la complessiva azione dell'amministrazione a rilievi in termini di coerenza e razionalità delle scelte adottate. La proroga è dunque una scelta inevitabile, per certi aspetti obbligata, fondata su valutazioni squisitamente, vorrei dire meramente, tecniche. Per quanto attiene più specificamente ai profili di carattere sanitario, segnalo che il comitato tecnico-scientifico che è stato interpellato dal Ministro della salute in merito all'opportunità di conservare le misure contenitive precauzionali adottate con la normativa emergenziale, ha reso, in data 24 luglio, un parere che contiene alcune considerazioni a mio avviso risolutive circa la necessità della proroga dello stato di emergenza. In primo luogo, il comitato rileva che, sebbene la curva dei contagi, così come l'impatto sul Sistema sanitario nazionale, si siano significativamente ridotti rispetto alla fase più acuta dell'infezione e questo è un dato positivo che dobbiamo tutti sottolineare perché ci rinfranca e ci induce a ripristinare quanto più possibile le pregresse condizioni di vita economica, sociale e culturale -, i numeri registrati documentano che il virus continua a circolare nel Paese, dando luogo, in alcune aree regionali, a focolai che al momento sono stati prontamente identificati e circoscritti. Il comitato segnala altresì che la situazione internazionale resta preoccupante - non dimentichiamo la questione internazionale - dal momento che si registrano in varie aree del mondo situazioni di contagio che non accennano a migliorare e che la situazione dei Paesi a noi vicini, addirittura confinanti - Francia, Paesi balcanici e Spagna - impone un atteggiamento di attenta vigilanza per evitare che la ripresa dei contagi interessi anche l'Italia. È lo stesso comitato tecnico-scientifico a sottolineare, infine, nel suo parere quanto ricordato poc'anzi: dopo la pausa estiva, nel mese di settembre dovrà essere garantita la ripresa dell'attività didattica frontale nelle scuole che interesserà complessivamente più di dieci milioni di persone. Le considerazioni espresse dal comitato rafforzano, dunque, con argomentazioni basate su evidenze scientifiche, le ragioni a fondamento della scelta di una proroga dello stato di emergenza e gli effetti anche di chiara utilità che essa è suscettibile di produrre. Lo ribadisco a beneficio della massima trasparenza: con questa decisione perseguiamo l'obiettivo di garantire continuità operativa alle strutture e agli organismi che stanno operando per il graduale ritorno alla normalità e che continuano a svolgere,

insieme - fortemente ridimensionata nella sua portata, non si è ancora esaurita. Con questa decisione consentiamo di prorogare gli effetti di misure necessarie la cui efficacia sarebbe compromessa in caso di cessazione dello stato di emergenza. Con questa decisione, infine, in base al principio di precauzione, in corrispondenza dei criteri che ci hanno sempre guidato sin qui di adeguatezza e proporzionalità, ci predisponiamo a mantenere un cauto livello di guardia, potendo così intervenire con speditezza ove mai dovessimo registrare un peggioramento della situazione. Ho letto tante cose e il dibattito pubblico, lo sappiamo, è molto vivace. Vi posso assicurare che da parte del Governo, mia personale e di tutti i Ministri, non vi è nessuna intenzione di drammatizzare, né di alimentare paure ingiustificate nella popolazione. La scelta di prorogare lo stato di emergenza non è affatto riconducibile alla volontà di creare una ingiustificata situazione di allarme, tutt'altro. Con la proroga dello stato di emergenza continueremo a mantenere in efficienza quel complesso di misure e iniziative organizzative, operative e funzionali che rendono il nostro Paese ben più sicuro, a beneficio dei cittadini italiani, ma anche dei turisti che volessero visitarlo. Lo testimonia l'indirizzo che ho voluto imprimere fin dalla conferenza stampa del 18 maggio, nella quale ho lanciato la fase 2. Da quel momento e in misura sempre più determinata ho sempre trasmesso - e sfido chiunque a dire il contrario - insieme ai Ministri segnali di massima fiducia, anche compiendo scelte risolute che, con un certo anticipo rispetto ai tempi inizialmente prefigurati, hanno favorito la ripresa della vita sociale e l'avvio in sicurezza delle attività economiche e commerciali. Dobbiamo correre; adesso dobbiamo procedere speditamente. Né la scelta di prorogare lo stato di emergenza può ritenersi lesiva della nostra immagine all'estero, in quanto suscettibile di alimentare la convinzione che l'Italia non sia ancora un Paese sicuro per turisti e lavoratori. Non vi è affatto questo rischio; anzi, come ho già detto, è vero il contrario: noi garantiamo un Paese più sicuro per tutti. L'Italia, alla quale tutti riconoscono il merito di aver affrontato molto bene la fase più acuta dell'emergenza, è attualmente da tutti vista come un Paese sicuro in grado di affrontare, proprio grazie alle necessarie precauzioni e a rigorose misure di monitoraggio e di prevenzione, la piena ripresa in sicurezza della vita sociale ed economica. Mi permetto di osservare - ma lo dico davvero con tono sommesso che anche questo dibattito parlamentare dovrebbe attenersi ai profili tecnici e giuridici della decisione, perché proprio un'impropria drammatizzazione del significato e degli effetti della proroga dello stato di emergenza - questa sì - sarebbe suscettibile di creare un potenziale nocumento all'immagine del Paese all'estero.

Vengo all'argomentazione che può apparire più insidiosa. Alla decisione di prorogare lo stato di emergenza sono stati attribuiti significati di ogni tipo, fino a prefigurare si è trattato, per carità, di voci isolate - la volontà di ricorrere a questo strumento al solo scopo di preservare, in capo al Governo o al Presidente del Consiglio, poteri *extra ordinem* suscettibili di alterare, tanto più se esercitati in assenza dei legittimi presupposti, l'ordinaria dialettica democratica, finanche il rapporto tra potere esecutivo e potere legislativo. È stata finanche sostenuta la paradossale tesi giuridica secondo cui sarebbe stato più opportuno procedere con ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge istitutiva del Sistema sanitario nazionale (la legge n. 833 del 1978), ritenendo addirittura che il ricorso a questo strumento fosse più garantista (semplici ordinanze del singolo Ministro) e più rispettoso dei presidi democratici rispetto al percorso da noi seguito che, come sapete, ha comportato l'adozione di norme di rango primario, attraverso lo strumento del decreto-legge, e conseguentemente anche l'emanazione di decreti del Presidente del Consiglio che, solo se considerate il procedimento di formazione ormai noto anche a tutti i cittadini, sono assistiti da numerose garanzie, ben superiori a quelle che assistono le ordinanze contingibili e urgenti, anche sotto il profilo della condivisione delle scelte, essendo previsto nel caso dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri il coinvolgimento dei Ministri e delle Regioni, come pure l'obbligo, che poi è stato introdotto specificamente dal decreto-legge n. 19 del 2020, di informare preventivamente le Camere. le Camere. Questa accusa si fonda su un evidente equivoco. Contrariamente a quanto spesso si sente dire, la proroga dello stato di emergenza non incide sul potere del Governo e del Presidente del Consiglio di emanare decreti. Lo stato di emergenza è il presupposto di fatto, ma non la fonte di legittimazione formale che si rinviene, invece, nella normativa introdotta da fonte di rango primario. Il potere, in particolare, di adottare ed emanare DPCM è al momento correlato alla data del 31 luglio, termine di cessazione dello stato di emergenza, non in ragione di una formale connessione tra i DPCM e lo stato di emergenza, ma perché questo espressamente prevede la fonte di rango primario legittimante, la quale avrebbe anche potuto disporre diversamente. In altre parole, qualora il Consiglio dei ministri adottasse la delibera di proroga dello stato di emergenza, non per questo il Presidente del Consiglio sarebbe autorizzato ad emanare DPCM. Il potere del Presidente del Consiglio dei ministri non deriva dalla dichiarazione dello stato di emergenza, né dunque si protrarrebbe per effetto della sua proroga, ma si radica - ripeto - nella normativa di rango primario. La dichiarazione dello stato d'emergenza costituisce certamente presupposto di fatto, il requisito sostanziale, ma non potrebbe di per sé in alcun modo legittimare l'adozione dei DPCM, se non fosse affiancata da una fonte - ripeto - di rango primario abilitante. Dunque, per poter continuare a essere esercitato dopo il 31 luglio, quel potere richiederà, comunque, un ulteriore intervento normativo, ovvero un nuovo decreto-legge che sarà sottoposto all'esame parlamentare per la sua conversione in legge. Con quel decreto dovranno, evidentemente, essere differiti i termini contenuti nei decreti-legge nn. 19 e 33, coerentemente con il termine prorogato dello stato di emergenza. Con successivi DPCM, poi, sempre in base ai principi di precauzione adeguatezza e proporzionalità, potranno essere confermate quelle misure precauzionali minime che ci stanno consentendo di convivere con il virus nella prospettiva di un pieno, benché graduale, ritorno alla normalità. In ogni caso, la mia presenza qui dimostra la massima disponibilità del Governo ad interloquire con il Parlamento, a tenere conto delle indicazioni che perverranno dalle Camere con riferimento alla scelta di prorogare lo stato di emergenza. Nel corso del Consiglio dei ministri che si è concluso questa mattina abbiamo inserito all'ordine del giorno una mera informativa. Non abbiamo adottato ancora nessuna decisione, per rispetto a questo dibattito che si sta sviluppando. però, dalla necessità di prorogare lo stato di emergenza, dopo aver esaminato in dettaglio tutte le implicazioni e i pareri acquisiti (ce n'è anche uno della dell'Avvocatura dello Stato), è emerso l'indirizzo di limitarne l'estensione temporale al prossimo mese di ottobre. Ricordo che lo stato d'emergenza fu dichiarato al Consiglio dei ministri, come ho detto all'inizio, il 31 gennaio, al verificarsi dei primi casi isolati di Covid-19 registrati all'interno di un gruppo di turisti cinesi che erano presenti a Roma. Peraltro, il Consiglio dei ministri assunse quella decisione dopo che, il 30 gennaio, l'Organizzazione mondiale della sanità aveva adottato la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per Covid-19. Sottolineo che questa decisione dell'Organizzazione mondiale della sanità è stata confermata il primo maggio. Mi rivolgo, dunque, alle forze di maggioranza, ma mi rivolgo anche alle forze di opposizione. Su queste questioni, io non credo si debba ragionare per schieramenti precostituiti o in base a logiche oppositive. Alla luce delle considerazioni svolte e dei dati obiettivi a disposizione - insisto su questo occorre essere consapevoli che la cessazione al 31 luglio dello stato d'emergenza determinerebbe l'arresto di tutto il sistema di protezione e di prevenzione costruito in questi difficili in questi difficili mesi, nell'interesse della collettività, a tutela di beni, quali la vita e la salute, che, sotto il profilo assiologico, sono al vertice della gerarchia dei valori costituzionali in quanto precondizione per il godimento di tutti gli altri diritti. Si è trattato di scelte difficili, che hanno comportato sacrifici, ma che ci hanno permesso di superare con successo le fasi più acute dell'emergenza. Sono scelte che il Governo ha sempre condiviso con il Parlamento, presentandosi davanti alle Camere, alla vigilia di ogni decisione. Resto quindi fiducioso che anche in questa occasione possa maturare qui, in quest'Aula, con consapevolezza e piena assunzione di responsabilità, una convergente valutazione positiva su questo decisivo passaggio, da cui discendono rilevanti conseguenze per l'intera comunità nazionale.

*(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci tengo ad iniziare questo intervento, invitando tutti a mantenere comportamenti responsabili e prudenti, perché il virus non è sparito e non è meno contagioso, prova ne sia la situazione in Belgio, ove hanno dovuto inasprire le misure di contenimento, a fronte di casi giornalieri più che triplicati nelle ultime tre settimane. Lo dico perché oggi intervengo in Aula all'indomani di un fatto, a mio avviso, gravissimo. Ieri, proprio qui, nel Senato della Repubblica, c'è stato chi ha rifiutato di indossare la mascherina: mi riferisco al senatore Salvini. Il senatore Salvini, forte di un 12 per cento scarso di presenze in quest'Aula, si è presentato qui, nel palazzo della seconda istituzione della Repubblica italiana *(Commenti)* per fare un atto di propaganda becero e senza senso. Viene qui per mandare un messaggio ai cittadini italiani, privo di qualsiasi fondamento scientifico. *(Proteste)*. Viene qui ad incitare le persone a non indossare la mascherina contravvenendo alle norme e alle regole di buon senso, che devono essere eseguite, per evitare che i contagi tornino a salire. Oggi, in Italia, vige l'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi pubblici al chiuso e vige quest'obbligo per delle ragioni ben precise. A quanto pare, pensare che i parlamentari lombardi conoscano la realtà dei loro territori e abbiano particolare sensibilità su cosa abbia significato per gli italiani il Covid-19 è mera chimera *(Commenti)*, ma, d'altronde, come dimenticare che era proprio il *leader* della Lega, a fine febbraio, a chiedere di aprire tutto e di far ripartire l'Italia. Fortunatamente c'è chi non ha ascoltato queste eresie ed è solo grazie a questo Governo se siamo riusciti a limitare i contagi da Covid-19. Questo però non vuol dire essere autorizzati a dimenticare quanto è successo negli ultimi sei mesi: i 246.286 casi in Italia, i 35.112 decessi, di cui 16.801 nella sua Regione. Non vuol dire essere autorizzati a dimenticare i mezzi militari carichi di feretri, che uscivano da Bergamo, gli accorati appelli degli operatori sanitari, stremati, che ancora combattono in prima linea. In queste situazioni, l'irresponsabilità non può essere perdonata. Mentre in Lombardia si moltiplicano le indagini della magistratura su quanto fatto dal governatore della Lega Attilio Fontana, anziché invitare a fare attenzione, in spregio di tutto e di tutti, c'è chi si permette di scherzare, dicendo che è giusto dare la mano a tutti e che la mascherina non serve. Purtroppo temo che ci siano ben poche parole per descrivere questi comportamenti. *(Commenti. Richiami del Presidente).*

Il professor Massimo Galli, infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano, ordinario di malattie infettive dell'università degli studi di Milano: «Penso che tutto quello che è stato detto non abbia alcuna base dal punto di vista scientifico: è un messaggio inadeguato, quello che viene lanciato, con elementi di evidente pericolosità». Il professor Fabrizio Pregliasco, virologo dell'università di Milano,

debba diventare un po' come gli occhiali da sole, da portare con noi e usare quando serve. Ovvero nei luoghi chiusi, affollati e all'aperto quando non si può rispettare il distanziamento». *(Commenti).* D'altronde purtroppo di questi atteggiamenti irresponsabili è pieno il mondo. Vogliamo parlare di Trump e di Bolsonaro? E infatti vediamo i drammatici risultati di gestioni politiche irresponsabili e cieche. Gli Stati Uniti e il Brasile sono in ginocchio per il Covid-19. In Italia fortunatamente a guidare il Governo non c'è la Lega, altrimenti non oso nemmeno immaginare che situazione vivremmo oggi. Grazie alle scelte coraggiose e responsabili di questo Governo, elogiate dalla comunità scientifica mondiale, a partire dall'Organizzazione mondiale della sanità, abbiamo rallentato i contagi, ma il virus c'è ancora e per questo non solo bisogna indossare la mascherina e mantenere le distanze di sicurezza, ma anche tenere alta la guardia, per esempio - e vengo a quanto stiamo discutendo in quest'Assemblea - prorogando lo stato di emergenza. Capisco che, se partiamo dall'assunto che il virus non c'è più, nemmeno la proroga dello stato di emergenza risulta necessaria. Ma è una menzogna, purtroppo. Non possiamo permetterci errori, non possiamo permetterci una seconda ondata, con quello che ne conseguirebbe. Dobbiamo fare tutto il possibile affinché questo non avvenga. Prorogare lo stato di emergenza è una di queste cose e far finta di niente, che non sia successo niente o, peggio, forzare la mano dicendo che ora è tutto finito è un atteggiamento che, lo ripeto, non ci possiamo permettere. Così come non ci possiamo permettere che i cittadini, per colpa di una becera propaganda elettorale, pensino che prorogare lo stato di emergenza si traduca in un nuovo *lockdown*. È vero il contrario: prorogare lo stato di emergenza, dare a questo Governo la possibilità di agire con tempestività è l'unico modo per prevenire che nuovi focolai possano espandersi tanto da metterci di nuovo in difficoltà. Penso, ad esempio, al blocco dei voli dai Paesi che hanno ancora migliaia di contagi. Eppure abbiamo esempi qui vicino di cosa può succedere.

per raccontare menzogne sull'uso della mascherina, per non prorogare lo stato di emergenza dando al Governo la possibilità di agire per tempo, facendo finta che il virus è stato sconfitto e facendo propaganda elettorale, sfruttando timori, anche legittimi, ai lavoratori tutti quando ci avrete riportato in una situazione grave? Come spieghereste che, per paura e banale leggerezza, il numero di decessi sia tornato a salire? Come fareste? Come il vostro governatore leghista Fontana che, pur di non assumersi la responsabilità, ha dato la colpa a tutti di quanto accaduto in Lombardia senza nemmeno scusarsi per quella drammatica ordinanza che mandò i casi di Covid-19 nelle RSA,

Senatrice Pirro, le vorrei dire che, sull'episodio di ieri, cui lei ha fatto riferimento, i senatori Questori stanno facendo un'istruttoria;

Colleghi, vi pregherei di stare ognuno al proprio posto perché c'è il problema - è vero - delle mascherine, ma c'è anche il problema degli assembramenti. occupa il posto che i senatori Questori gli hanno attribuito, possiamo condurre una discussione in maniera un po' più tranquilla.

Avevo scorto un po' di preoccupazione nell'intervento del Presidente del Consiglio, che ci ha ripetuto più volte che l'eventuale non conferma dello stato di emergenza farebbe in qualche modo decadere tutta una serie di misure. Ce lo ha ripetuto all'inizio e a metà dell'intervento, e giustamente, rivolgendosi alla maggioranza e anche all'opposizione, lo ha precisato al termine dell'intervento. Ha voluto, quindi, ricordarci nuovamente che la mancata proroga dello stato di emergenza farebbe decadere una serie di misure straordinarie che sono state emanate nel frattempo. Presidente Conte, devo dire che apprezzo sempre il lavoro di coloro i quali si interessano in particolare della salute pubblica, e ammetto che l'Italia, come lei ha ricordato, si è mossa forse meglio di qualche Paese europeo in ambito sanitario per quanto riguarda, appunto, l'attenzione alla diffusione del virus. Tuttavia, non è passato inosservato che, rispetto a tutto ciò che oggi è obbligatorio nella fase 3 già nella fase 2) ovvero l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, il distanziamento tra persone,

isolati, ma che è necessario prestare la giusta attenzione. Io credo che il problema sia *ab origine* della quando l'Italia non è stata pronta nell'evitare un *lockdown* obbligatorio per tutti, cosa che non è avvenuta anche in gran parte degli Stati europei,

una visione; vuoi che lo stato di emergenza era arrivato fra capo e collo, vuoi che l'incremento dei casi era in crescita esponenziale. Va tutto bene, il problema è che non eravamo pronti non eravamo pronti e oggi andare nuovamente a prorogare lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, quando lei - e l'ho apprezzato - ha voluto precisare

non voglio ricordare che è un fatto doveroso per il Governo presentarsi in Parlamento, in particolare in questo momento - se ci sono delle cose che non ci ha detto, signor Presidente infatti con le premesse fatte e con l'opportunità del Governo di emanare anche provvedimenti di urgenza, con una semplice convocazione di due Ministri oltre a lei, anzi credo uno, visto che il Consiglio dei ministri non è soggetto al numero legale, lei può emanare decreti-legge ad ogni piè sospinto. Io sono alla prima legislatura, come lei, anche se lei è in una posizione diversa dalla mia. Criticavo anche i Governi di centro-destra che sfornavano decreti. Devo dire che, pandemia o non pandemia, in questi due anni di decreti-legge ne abbiamo visti ogni giorno. E allora per quale motivo non possiamo individuare tutti i provvedimenti che andrebbero ad essere terminati relativamente al periodo di emergenza all'interno di un decreto-legge che li mantenga in vigore per eventuali necessità? Perché non lo facciamo? Non ci meravigliamo poi se si rincorrono le voci che questa ulteriore proroga potrebbe in qualche modo mettere in sicurezza la sua maggioranza, oppure la durata del Governo. Qualche Qualche malalingua potrebbe ancora pensare che essendo convocate le elezioni amministrative regionali e il *referendum* per il 20 e 21 settembre, vuoi vedere che essendo poi prorogato anche lo stato di emergenza al 31 ottobre, non ci potrebbe essere anche

però che queste problematiche non sono soltanto il pensiero del senatore Mallegni o del Gruppo Forza Italia, ma albergano in tutto l'arco costituzionale. Lei oggi viene a chiedere al Parlamento un atto di responsabilità; il Parlamento l'atto di responsabilità lo ha fatto dal primo momento in cui si è reso disponibile, in particolare nei Gruppi a dare credito al suo Governo e domani ci sarà un atto sullo scostamento di bilancio, che ulteriormente dovrà rendere responsabile, in particolare questo ramo del Parlamento, nell'offrire al Governo e all'Italia l'opportunità di andare a recuperare ulteriori risorse, perché le risorse sono mancate. Io, che faccio l'imprenditore nel settore turistico, le do la mia parola d'onore: ci sono nostri dipendenti e collaboratori che non hanno avuto la fortuna di essere reimpiegati (perché il calo di lavoro oscilla dal 50 al 75 per cento in quel settore), i quali ancora non hanno ricevuto la cassa integrazione.

a coloro i quali devono spendere e investire nel nostro Paese per tentare di sostenere il prodotto interno lordo, di continuare a farlo, però con la spada di Damocle di un ulteriore periodo di emergenza che non rende nessuno sereno. Gli investimenti? Non possiamo chiedere investimenti ulteriori. La spesa? Non possiamo chiedere spesa ulteriore. Delle due, l'una: se lei ci chiede questo impegno - e lo fa con responsabilità e senso del dovere - noi le vogliamo credere,

A fronte di questa richiesta di responsabilità deve esserci la responsabilità anche di tutti gli attori in campo. Lei ci deve garantire questo e deve fare in modo che chi opera al di fuori del Governo, ma ha la responsabilità nei confronti degli italiani, agisca in modo consequenziale. Solo in questo caso lei avrà il nostro consenso.

lei è stato molto chiaro e circostanziato, come le compete. Per definire il suo *modus operandi* voglio usare alcuni termini che hanno guidato ogni suo passo: equilibrio, forza, tenacia e cautela. Ricordo anche il suo approccio filologico, quello che lei sintetizzò con il termine «umanesimo», facendo riferimento alla nostra più grande storia: l'umanesimo quale rinascita europea dopo decenni bui. È però il termine «equilibrio» quello che ritengo più importante e caratterizzante la sua azione, quell'equilibrio che in tutti i fenomeni naturali è la risultante di grandi forze, così come nascono spesso le nostre più difficili decisioni, esito di contrapposte riflessioni e considerazioni. Nessuno nel dicembre 2019, quando la commissione sanitaria di Wuhan segnalava all'Organizzazione mondiale della sanità un *cluster* di casi di polmonite a eziologia ignota, poteva minimamente immaginare cosa sarebbe successo in Italia di lì a poco, dovuto registrare, a oggi, in pochi mesi, più di 35.000 decessi. Non avremmo mai potuto immaginare 600.000 decessi e 15 milioni di casi confermati nel mondo Eravamo consapevoli di essere stati chiamati a guidare il nostro Paese in una difficile situazione, ma non ci si aspettava l'epocale tormenta che stiamo attraversando. Chi è un po' più maturo ricorda ancora i racconti dei nostri avi, quelli dell'influenza spagnola. Oggi i nostri stili di vita sono assai diversi da allora, ma nei confronti degli attacchi virali il risultato, purtroppo, non cambia. Siamo stati chiamati a gestire una delle situazioni più difficili dal Dopoguerra a oggi. Continua ad essere utile e indispensabile ogni azione di prevenzione, che tutti dobbiamo continuare a mettere in atto.

ma in questa singolar tenzone l'umanità sta tutta da una parte e questo dovrebbe essere chiaro a tutti. Vado un po' fuori tema, ma oso. Un sano scatto d'orgoglio dovrebbe oggi guidare anche quelle riforme strutturali di cui si parla da diversi lustri, perché l'Italia possa intraprendere un nuovo corso. I prossimi mesi non saranno facili per nessuno, ma la politica potrà riconquistare un ruolo certamente più significativo: da una parte sarà chiamata a incidere nella tutela della salute di tutti, donne e uomini di questa Europa, dall'altra dovrà tutelare il lavoro di ognuno e le aziende che lo creano. In questa partita la finanza, che è stata finanche chiamata creativa, dovrà cedere il passo. Ripeto che tutti dovremo fare la nostra parte e - uso un termine non più di moda - tutti dovremo fare il nostro dovere. Mi preme aggiungere che occorrerà riflettere assai sugli investimenti che saranno programmati. Penso agli investimenti in infrastrutture capaci non solo di fare da volano momentaneo, ma utili soprattutto a creare sviluppo futuro. Accenno sinteticamente, a titolo esemplificativo, a un piano di manutenzione straordinario di ogni infrastruttura. In preda al costume dell'usa e getta, sempre più dominante, e dell'utile economico, fattore prioritario spesso unico, abbiamo abbandonato ormai il concetto stesso del termine manutenzione, quella già definita da tanti testi normativi semplicemente ordinaria. un piano di investimenti per la nostra terra, nel nostro settore dell'agroalimentare, *brand* italiano di prestigio planetario. Penso a nuove reti di irrigazione, per aiutare le nostre aziende agricole a risparmiare e tutelare la preziosa risorsa idrica. Penso alla tutela del *mare nostrum*, dei nostri paesaggi e di ogni vestigia che i nostri avi ci hanno lasciato, quali ricchi eredi che siamo, spesso anche inconsapevoli. Si tratta di risorse tutte uniche e non delocalizzabili. Sarà la bellezza a salvare il mondo, se è accompagnata dal buon senso; e il popolo italiano ha sempre dimostrato di averne tanto di buon senso, anche in questa fase. Occorrerà avere fiducia, quella verso il prossimo, capace di far sentire un più autentico senso anche della cosa pubblica. Concludo con l'augurio che mi piace pronunciare nella vita di tutti i giorni: buon lavoro, signor Presidente, e buon lavoro a tutti noi, anche nella difficile situazione di emergenza.

presidente Conte, innanzitutto lei viene a chiederci di votare uno stato di emergenza in un momento in cui, nel nostro Paese, sono quattro giorni che non ci sono decessi e in cinque Regioni non c'è nessun nuovo caso di Covid. Sembra un po' inopportuno sui tempi. Viene a chiederci lo stato di emergenza in un Parlamento dove impera la paura, ma non paura da mascherina: paura da elezioni. *(Applausi)*. Il partito della cadrega ha paura di andare a votare e quindi le voterebbe qualsiasi cosa in questo momento, signor Presidente. a proporre uno stato di emergenza per zittire gli italiani, come sta provando a fare questa maggioranza con il sottoscritto, perché sto provando a parlare e stanno già iniziando a protestare. Uno stato di emergenza non previsto dalla Costituzione, signor Presidente, perché la Costituzione non prevede lo stato di emergenza. Ricordo che durante gli studi universitari il mio professore di diritto costituzionale, il professor Bettinelli, mi disse una volta: «Se vuoi avere l'arroganza e l'autorevolezza di rappresentare gli italiani, devi conoscere la Costituzione ci dice esattamente che lo stato di emergenza non è previsto; ahimè per lei non siamo in Francia, ahimè per lei non siamo in altri Paesi europei, ma siamo in Italia *(Applausi)*, dove la Costituzione le permette, in casi di necessità e di urgenza, di utilizzare lo strumento del decreto-legge. Quindi, purtroppo, lei va contro la Costituzione della Repubblica Italiana. *(Applausi)*. Cosa ha prodotto lo stato d'emergenza finora?

italiani *(Applausi)*, perché ieri l'Istat ci ha detto che entro il 31 dicembre si stima che un milione di cittadini italiani sarà a casa senza lavoro; e non lo dicono il cattivone Centinaio della Lega o quelli che non propongono niente, ma l'Istat,

Il problema è che il ministro De Micheli il traffico non lo trova, perché forse gira in elicottero. *(Applausi).* Serve al ministro Bellanova, che con la pagliacciata del pianto

che è tanto, signor Presidente. Zero idee e zero progetti, solo promesse e prese in giro. Tutte le associazioni del turismo, nessuna esclusa, stanno contestando il ministro Franceschini: il problema è che tutta questa gente vorrebbe scendere in piazza, ma non può, perché, visto e considerato che c'è lo stato d'emergenza, non può protestare, signor Presidente del Consiglio, e non può farle capire cosa pensa realmente di lei. Oppure serve a lei, signor Presidente, per tenere al guinzaglio il Parlamento e impedire agli italiani di scendere in piazza e farle capire, come le ho detto, che il suo tempo finalmente è finito. Il problema è che sembriamo quegli Stati autoritari in cui nessuno deve permettersi di criticare il manovratore: nessuno deve far notare il grande imbroglio di questi mesi, il grande gioco dell'oca che aveva un solo obiettivo, la visibilità del *Premier*. Prima fase: conferenze stampa per far credere agli italiani che la maggioranza fosse forte e coesa e che ce l'avrebbe fatta da sola. dell'oca: stava per arrivare al via, ma decide di fare una nuova conferenza stampa, per far credere che il Governo avrebbe teso la mano alle opposizioni; una bufala smentita in queste Aule parlamentari. Terzo gioco dell'oca, terza fase: conferenza stampa per far credere al popolo che saremmo usciti dall'emergenza grazie ai saggi nominati dal Governo. Non si sa cosa stiano facendo e cos'abbiano fatto. Quarta fase: imbarazzante sceneggiata degli stati generali a Villa Pamphili, con tanto di conferenza stampa, per riempire la testa degli italiani. E ora, visto che le precedenti non hanno portato a niente, perché ormai la gente si chiede cos'avete intenzione di fare adesso, arriva la quinta fase, in cui il nostro supereroe veste i panni dello statista internazionale che impone all'Europa le sue idee e porta a casa tanti soldi. Quando non si sa, ma porterà a casa tanti soldi. Nel frattempo, in Italia le aziende chiudono e le famiglie sono sempre più in difficoltà. Lei lo sa, signor Presidente, che, da una indagine che è stata fatta dalla grande distribuzione, lo scontrino medio è sempre più basso? E lo scontrino medio sempre più basso nella grande distribuzione vuol dire che le famiglie non hanno più soldi,

Che immagini ci restano di questi mesi di Covid, oltre a quelle delle bare di Bergamo, che ricordiamo tutti e non c'è bisogno che la collega le ricordi e ci ricordi cosa è successo a Bergamo? Ci rimane l'immagine di questi giorni e delle scorse settimane: le Forze dell'ordine che rincorrono una persona che in una spiaggia stava prendendo il sole in un momento del *lockdown*. Ridicolo, una persona rincorsa da tutte le Forze dell'ordine. Ci rimane l'immagine degli alpini a Ventimiglia in assetto antisommossa - avevano persino il mitra - in spiaggia per mantenere la distanza di sicurezza. Mentre si andava dai turisti a far mantenere la distanza di sicurezza, ci rimangono l'immagine, le foto e le videoriprese dei migranti che scappano dai centri di accoglienza.

i migranti vestiti da turisti - che vengono accolti, con tanto di telefonino, sigaretta in bocca e il barboncino al guinzaglio. *(Applausi).* Siete imbarazzanti, questi sono i turisti che piacciono a voi. Vi piacciono talmente tanto, questi turisti, che avete bloccato gli accessi dei turisti altospendenti, quelli veri, che avrebbero portato soldi nel nostro Paese, e invece in zone turistiche, come ad esempio a Fiuggi (in un bell'hotel di Fiuggi), ci sono sessanta migranti. Questo è il modo in cui trattate le aree termali del nostro Paese.

che ha dato la linea che lei deve seguire. Tre regole: uso delle mascherine, distanza di un metro, frequente lavaggio di mani. Non serve lo stato di emergenza; gliel'ha detto il suo Ministro cosa bisogna fare; non serve lo stato di emergenza per permetterle di mantenere la cadrega. I pieni poteri - perché questi sono i pieni poteri - senza passare dalle urne non fermano il Covid, ma servono solo per farvi stare comodi sulla cadrega. un auspicio personale. I pieni poteri fino al 31 ottobre, il giorno del mio compleanno. Farò dunque di tutto per farmi un regalo: la caduta di questo Governo,

Per cortesia, ci sono i senatori Questori che in quest'Aula mantengono l'ordine.

Dai banchi della Lega è emerso in maniera chiarissima - io l'ho sentito e sono dalla parte opposta - la definizione della senatrice Pirro «oca parlante». Lei non può permettere che questo accada. Senatore Bressa, siccome quando uno parla fuori dal microfono non arriva tutto alla Presidenza,

della Presidenza non si sente nulla, se uno parla fuori dal microfono. Spesso vi agitate, ma qui non arrivano le vostre proteste.

signor Presidente del Consiglio dei ministri, signori rappresentanti del Governo, gentili colleghe e colleghi tutti, prendo la parola in quest'Aula per rispondere a talune dichiarazioni e anche a taluni comportamenti di alcuni esponenti delle forze di opposizione riguardo alla decisione assunta dal Governo con la richiesta di proroga dello stato di emergenza, richiesta che ritengo assolutamente coerente con lo stato delle attuali contingenze e improntata a principi di precauzione, di prudenza e di prioritaria tutela della vita e della salute dei cittadini. È bene precisare e ribadire che l'epidemia da Covid-19 non può considerarsi superata e archiviata, questo è risaputo. Siamo certamente lontani dai numeri dei mesi scorsi e, anche se in alcune Regioni - com'è stato detto non ci sono stati nuovi casi, è anche vero che l'indice Rt in altre Regioni è ancora superiore all'unità. È vero, comunque, che il *trend* epidemiologico in Italia oggi appare piuttosto rassicurante questo grazie ai corretti e adeguati provvedimenti adottati dal Governo, motivo per cui al momento non vi sono particolari criticità. tuttavia non deve assolutamente indurci ad abbassare la guardia e non vuol dire che questo Coronavirus sia stato debellato e che sia un lontano nemico, tutt'altro; esso è sempre presente e vicino e lo dimostrano i tanti focolai che si registrano anche oggi in molte Regioni italiane. Il virus sta ancora circolando e ciò si può paragonare alla situazione di un incendio che è stato domato, ma che non è ancora del tutto spento perché, come fuoco sotto la cenere, nuovi *cluster* continuano a emergere, interessando prevalentemente oggi individui più giovani rispetto a quelli colpiti nei mesi precedenti, così come anche nuovi *cluster* si costituiscono per via dei cosiddetti casi di importazione, i quali ultimi necessitano di un'ancora più stringente e costante attività di controllo e prevenzione da parte delle istituzioni, con particolare riguardo al fenomeno migratorio. Quanto accade in altre parti del mondo mostra che il virus è ovunque ancora presente e che, se non viene tempestivamente arginato, l'infezione rischia di crescere e accelerare. Basti pensare alla drammatica situazione di alcuni Paesi del Sud America, come il Brasile, con oltre un milione di casi o, ancora, ai 4,4 milioni di individui contagiati negli Stati Uniti o al milione e mezzo di infetti in India. Proprio la difficoltà di tenere sotto controllo la pandemia ha portato all'esclusione degli Stati Uniti, oltre che della Russia e del Brasile, dalla lista dei Paesi i cui cittadini potranno rientrare nell'Unione europea a partire dal 1° luglio, cioè da quando sono state riaperte le frontiere esterne alla stessa UE. Hans Kluge, direttore regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità, ha espresso la sua preoccupazione: «la scorsa settimana in Europa si è registrato un aumento dei casi settimanali di Covid-19 per la prima volta da mesi». In particolare in 11 Paesi, ha dichiarato: «la trasmissione accelerata ha portato ad una ripresa molto significativa che, se non controllata, spingerebbe di nuovo i sistemi sanitari sull'orlo della crisi». In una nota alla stampa Kluge ha avvertito che dobbiamo prepararci all'autunno, quando Covid-19 potrebbe incontrare anche l'influenza stagionale, polmoniti e altre malattie, perché alla fine il virus circola ancora attivamente nelle nostre comunità e non esiste ancora alcun trattamento o vaccino efficace. Non dobbiamo farci trovare impreparati qualora il contagio dovesse risalire la curva nel prossimo autunno. La prudenza, il rispetto delle norme di igienizzazione e di distanza fisica, l'uso della mascherina sono da mantenere anche negli spazi aperti ed occorrerà ancora più prudenza al termine dell'estate, quando diminuiranno le occasioni per stare all'esterno ed aumenteranno le possibilità di vicinanza e di contatto fisico. Cautela, prudenza, rispetto delle norme per la tutela della nostra salute e della nostra vita devono essere le parole d'ordine. È anche ciò che dobbiamo a chi ha sacrificato la propria vita per proteggere quella degli altri, al personale medico e sanitario soprattutto, ma anche a tutti quei lavoratori e professionisti che si sono adoperati perché potessimo continuare ad usufruire dei beni di prima necessità durante il periodo del *lockdown*. Il fatto che in Paesi diversi ma con condizioni climatiche e di vita sociale molto simili al nostro come la Spagna e il Portogallo, il virus abbia rapidamente ripreso a circolare in queste ultime settimane, deve farci riflettere sulla facilità con la quale potremmo trovarci nuovamente in una condizione di emergenza, con la conseguente necessità di assumere tempestive ed adeguate decisioni. È indubbio che bisogna rafforzare il patto di collaborazione tra Governo e Parlamento, come lei giustamente sta facendo signor Presidente del Consiglio dei ministri, ma è anche altrettanto vero che bisogna fornire al Governo gli strumenti per prendere tempestivi ed appropriati provvedimenti nelle circostanze di una possibile e non escludibile ripresa dell'epidemia. Riteniamo giusto e doveroso sostenere un Governo che pone al centro delle proprie decisioni la tutela della vita e della salute dei cittadini. Questa linea di comportamento è ciò che ha permesso di salvare migliaia di vite umane ed è su questa linea del Governo che riteniamo giusto continuare. *(Applausi)*.

di come si stia affrontando, anche in quest'Aula, la grave situazione in cui versa il nostro Paese. Parliamo soprattutto della grave, gravissima situazione sociale, economica e produttiva che l'Italia paga più di altri Paesi. Vede, signor Presidente, la maggioranza viene condotta in maniera riluttante a questo provvedimento di proroga dello stato di emergenza, al punto tale che sino a questo momento hanno parlato tre esponenti del suo partito di riferimento, cioè dei 5 Stelle, e nessun altro della maggioranza, che ovviamente prenderà la parola in maniera stringata successivamente per confermare

e noi ne siamo rallegrati - nel giustificare lo stato di emergenza si richiamano alla scienza e ai vaccini, dopo aver negato per tanto tempo la validità della scienza e l'efficacia dei vaccini.

la piattaforma Rousseau e i *referendum* su ogni piccola decisione che avrebbero dovuto prendere, la sospensione delle regole democratiche e dei diritti dei cittadini per decreto del

ritiene doverosa questa concessione ci preoccupa per la sua postura nei confronti del Parlamento. Allo stesso modo ci preoccupa il fatto che lei dia indicazioni in Parlamento su come si deve svolgere il dibattito: scusi se glielo faccio notare, ma lei ha detto che il dibattito dovrebbe attenersi ai giudizi tecnici e solo a questo.

Io credo che questo debba preoccupare tutti, tanto più a fronte - glielo dico - della inconsapevolezza con cui affrontate

Consiglio dei ministri e cavilli giuridici per sospendere libertà costituzionali senza rendervi conto del fenomeno che abbiamo davanti e che avrebbe bisogno di altra consapevolezza, di altra responsabilità, di altra determinazione. Abbiamo avuto un'accelerazione della storia, che per esempio nel campo del lavoro e della società si è tradotta nel fatto che oggi tutti parlino e utilizzino lo *smart working,* con problemi di innovazione tecnologica e di espulsione dal mercato del lavoro:

ma nell'arco di anni, di decenni e che invece sono accadute l'arco di giorni. Si è assistito all'accelerazione di un fenomeno globale, il conflitto in atto tra la Cina e gli Stati Uniti, con l'India che si schiera con gli Stati Uniti contro la Cina, in un conflitto globale che sarebbe certamente avvenuto nell'arco dei prossimi anni (ce n'erano tutte le avvisaglie e solo voi non lo avete capito quando avete firmato il documento sulla nuova via della seta)

di come non vi rendiate conto di ciò che l'Italia dovrà affrontare di fronte alla crisi globale di cui noi siamo l'epicentro. Lo dimostra il fatto che ogni stima per l'Italia è ogni

Per cui oggi - o meglio, domani - noi avremo un altro scostamento di bilancio di altri 25 miliardi (e siamo già a 100 miliardi in più di indebitamento diretto) e stiamo prospettando un altro indebitamento nei confronti dell'Europa senza nel frattempo predisporre nulla.

Quanta consapevolezza c'era in quella classe dirigente, che non ha avuto bisogno di applicare uno stato di emergenza per fronteggiare una drammatica, quella sì, condizione di attacco al cuore del nostro Paese. Non la trovo in voi questa consapevolezza, questa responsabilità, questa statura. Non la trovo, purtroppo, in questo Senato e questo, davvero, è quello che ci preoccupa di più.

a quest'Assemblea non è di poco conto. La proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre non è un semplice passaggio formale. Si tratta di contemperare le libertà fondamentali, da un lato, e i diritti, come quello alla salute, dall'altro, con la necessità che l'azione del Governo sia mirata, veloce e tempestiva nel caso in cui dovesse esserci una recrudescenza del virus.

anche nell'emergenza, è fondamentale operare un bilanciamento fra la necessità che la decisione sia veloce ed efficace e il rispetto di quelle prerogative costituzionali che la Costituzione affida al Parlamento (ripeto, al Parlamento), che deve essere, sempre e comunque, centrale, perché è qui che si esprime la sovranità popolare. L'emergenza sanitaria ha messo in ginocchio il Paese, soprattutto il Nord. Abbiamo pianto 35.000 morti e l'immagine delle bare di Bergamo resterà per sempre indelebile nelle nostre menti. Oggi, però, l'emergenza sanitaria è conclusa. Certo, occorre rispettare le misure di sicurezza e di stanziamento, indossare le mascherine, ma le terapie intensive sono fortunatamente vuote e abbiamo anche imparato ad isolare in modo efficace i contagi. Al contrario, ci sono altre emergenze che rischiano di esplodere in autunno, prima di tutto quella economica. L'Europa ha fatto la sua parte con il *recovery fund*, ma ora occorre elaborare un piano preciso per aiutare il Paese a risollevarsi, sostenere le aziende in sofferenza, il settore del turismo e la manifattura, tutelare le nostre eccellenze, tutelare i nostri ristoratori, i commercianti. Dobbiamo, in sostanza, abbandonare l'assistenzialismo. A maggio sono state pagate più pensioni che stipendi. Un Paese che non interviene sul sostegno ai lavoratori è un Paese senza futuro. Basta, allora, con le casse integrazioni e puntiamo di più sulla decontribuzione, come ha fatto il *jobs act*. Investiamo in grandi opere ed eventi. Il Nord, che è stato particolarmente colpito dal virus, come sappiamo, ospiterà ad esempio le Olimpiadi invernali del 2026. Un evento che porterà certo tanti visitatori, ma anche infrastrutture che resteranno che resteranno alle Regioni interessate (Veneto, Lombardia e Trentino) e che contribuiranno a ridare respiro a queste Regioni, che sono le più colpite dal virus. Esiste poi un emergenza altrettanto pressante, lo dico prima di tutto da madre: quella educativa, che troppo spesso rischia di passare in secondo piano. La scuola, signor Presidente del Consiglio. Quando chiedemmo di riaprire le scuole a maggio, gli italiani ci presero per pazzi, però poi ci dettero ragione. Riaprire le scuole e consentire che le lezioni riprendano dal vivo a settembre è fondamentale per i nostri ragazzi. La scuola ha la funzione di formare i nostri figli e di renderli dei cittadini consapevoli. È grazie all'istruzione che si combatte la disparità sociale, eppure è un tema ancora troppo sottovalutato dalla politica. Come candidata presidente della Regione Veneto ho provato a coinvolgere in modo *bipartisan* gli altri candidati presidenti

Le famiglie, tutte le famiglie, hanno già pagato troppo in termini di sacrifici e difficoltà; i bambini e i ragazzi sono stati messi in una condizione di incertezza e di precarietà inaccettabili, per non parlare del fatto che, chiudendo le scuole, si impedisce loro, spesso, anche di praticare lo sport di base. Molte associazioni, infatti, utilizzano le palestre dei complessi scolastici. sport non è meno importante della formazione culturale, che va garantita ai nostri ragazzi. Allora dico: non nascondiamoci dietro la paura del contagio. Per ripartire occorre avere fiducia! Qualche tempo fa, dei pediatri inglesi hanno scritto una lettera aperta, che condivido in pieno, che evidenzia come tenere chiuse le scuole lascerà dei danni indelebili ai ragazzi. signor Presidente, è giusto prorogare lo stato di emergenza fino al 15 ottobre, ma chiediamo che ci sia un intervento immediato sulle scuole.

che le scuole, dopo essere state ferme per sei mesi, riaprano a settembre, per poi essere chiuse nuovamente, qualche giorno dopo, per stabilirvi i seggi elettorali. I nostri ragazzi e le nostre famiglie non possono essere ancora una volta destabilizzati. Per questo - e concludo - ho scritto al ministro Lamorgese, affinché siano individuati altri luoghi dove svolgere le votazioni. Ho chiesto che entro il 14 agosto sia realizzata una mappatura di questi luoghi ed entro fine agosto venga erogato il finanziamento ai Comuni per le spese afferenti alle nuove tessere elettorali e per l'informativa ai cittadini sulle nuove sedi. Come diceva Nelson Mandela, «l'istruzione è l'arma più potente che puoi utilizzare per cambiare il mondo». Signor Presidente, saremo al suo fianco, ma non si dimentichi dei nostri ragazzi e delle nostre famiglie.

Presidente, membri del Governo, colleghe e colleghi, signor Presidente del Consiglio, dico subito che, ad avviso del Partito Democratico, la proposta, che oggi ci viene rivolta, di una limitata proroga dello stato di emergenza è una decisione tecnicamente necessaria, per le ragioni che lei ha detto, e una decisione politicamente saggia, perché andare in questa direzione significa voler fare l'interesse dei cittadini. Fare l'interesse dei cittadini italiani e difendere il Paese dovrebbe essere sempre la nostra principale preoccupazione. Raramente alzo i toni, ma devo dire che quando, nell'intervento di un collega dell'opposizione, molto impostato sui toni del comizio, ho sentito che la ragione per cui si viene in Parlamento - ora in Senato e dopo alla Camera - a chiedere la proroga dello stato di emergenza è la ricerca di pieni poteri e di un modo per zittire il dissenso, ho provato sdegno, vero sdegno, perché non è possibile mettere le cose su questo piano. Vorrei dire al collega Centinaio, che ci ha deliziato con questa teoria, che forse sono le forze con cui lui va a braccetto in Europa che, nei loro Paesi, cercano di zittire il dissenso e cercano i pieni poteri. Non crediamo sia il caso di fare polemiche in una circostanza così grave, ma alcuni puntini sulle i vanno messi. Ritengo che, in una situazione come quella che ci troviamo di fronte, chi rappresenta le istituzioni abbia un dovere, come ha ricordato molto bene, in una sua dichiarazione stamane, il Ministro della sanità, che ringrazio per il suo lavoro e per la sua attenzione alle prerogative del Parlamento, che non è mai mancata: sulle regole essenziali - e sono ormai poche le regole essenziali che dobbiamo rispettare e vengono ricordate ogni giorno tutti dovremmo essere uniti. Specialmente chi rappresenta le istituzioni dovrebbe essere unito. Non è possibile che ci dividiamo proprio sull'essenziale e non è possibile che chi sta nelle istituzioni abbia sempre la tentazione di dare il cattivo esempio, di mettere in atto atteggiamenti diseducativi, di predicare cose che contrastano con le regole. Ieri in Senato non è avvenuta una bella cosa, perché non si avalla mai un convegno negazionista sul Covid-19 quando si è in una situazione come quella in cui siamo. *(Applausi)*. Chi sta nelle istituzioni dovrebbe essere unito, non soltanto nella difesa delle regole essenziali, ma anche nel raccomandare ai cittadini di non metterne in dubbio la fondatezza, nel rimproverare chi va in senso opposto e nel deplorare quelle immagini che purtroppo vediamo nei telegiornali e sui giornali, che mostrano assembramenti che non vanno bene, la mala *movida*, troppi giovani che sembrano prendere eccessivamente alla leggera il pericolo che corriamo e che mettono in campo comportamenti che devono essere stigmatizzati. Non bisogna lisciare il pelo di chi vuole buttarsi quello che abbiamo vissuto alle spalle, in nome di una irresponsabilità senza capo né coda. Dobbiamo essere estremamente severi. La riflessione che facciamo sullo stato di emergenza dovrebbe servire soprattutto a questo. Credo non sia convincente - voglio essere estremamente chiaro - l'argomento di chi dice che non dovremmo prorogare lo stato di emergenza perché non siamo più in emergenza. È un'affermazione sbagliata; è un'affermazione che non ha basi, perché non è affatto vero che siamo fuori dall'emergenza. Io credo che siamo in un periodo diverso dell'emergenza, in una fase meno acuta dell'emergenza, ma è innegabile che ancora oggi corriamo dei rischi, che ci pongono nella necessità di adoperare strumenti che non fanno parte dell'ordinarietà. È allora inutile giocare con le parole: se le istituzioni hanno bisogno di attivare strumenti che non fanno parte dell'ordinarietà, è giusto che propongano al Parlamento, confrontandosi con chi sta in Parlamento, un prolungamento dello stato di emergenza, che ci consenta di decidere adeguatamente e con la rapidità necessaria. Noi abbiamo un dovere nei confronti delle tantissime persone che ci hanno aiutato a fronteggiare

i pericoli e i rischi che l'Italia corre, ancora oggi, anche se i malati sono 12.000 e non più decine e decine di migliaia. Infatti i malati sono 16 milioni nel mondo abbiamo visto che, dove le istituzioni hanno preso decisioni sbagliate e hanno dato esempi sbagliati, la situazione tende ad andare fuori controllo. Noi non possiamo attuare suscettibili di far impennare la curva dei contagi, perché faremmo qualcosa di contrario agli interessi dei nostri concittadini e di molto pericoloso per la loro salute. nel dire che siamo in una fase differente dell'emergenza si dice una cosa che ha un peso e un significato preciso. Stiamo dicendo, cioè, che non siamo più nella condizione nella quale ci trovavamo a marzo, ad aprile o a maggio; quindi, anche il nostro stare nell'emergenza e il nostro decidere nell'emergenza devono avere caratteristiche tali da essere compatibili con la diversa fase che stiamo vivendo. Probabilmente abbiamo bisogno di provvedimenti che abbiano una dimensione temporale e territoriale più circoscritta, più mirata, meno indiscriminata. Abbiamo bisogno che la proporzionalità delle decisioni che assumiamo diventi veramente una delle grandi preoccupazioni che ci muovono nel decidere, nell'elaborare i provvedimenti, nello studiare quello che serve per fare tutto quanto è necessario in questo momento. Da questo punto di vista - e concludo - è davvero fondamentale il coinvolgimento del Parlamento. Credo che sia qualcosa di utile per il Governo, di prezioso per chi è chiamato a decidere in emergenza e fuori dall'ordinarietà, di doveroso nei confronti di un'istituzione che rappresenta il popolo italiano e che ha il diritto e il dovere di fornire contributi di riflessione e di proposta che arricchiscono chi li dà e - penso - anche chi li riceve.

Presidente Conte, Ministri, onorevoli colleghi, ci troviamo nuovamente qui, per l'ennesima volta, a

capire che effettivamente il Parlamento, questa sede, è il luogo del confronto, fermo restando che sappiamo che di quello che pensano e dicono le minoranze a lei poco importa. Se, poi, il dalla Lega, come un bambino dispettoso fa esattamente l'opposto di quanto le viene detto. per lei ma noi siamo con gli italiani; in questo luogo continueremo a dire la verità agli italiani e continueremo a dar voce a due verità, anche se scomode per lei. Lei ha deliberato lo stato di emergenza il 31 gennaio, in barba alla Costituzione italiana, perché, diversamente da quanto previsto nella Carta francese, in quella ungherese e in quella spagnola, nella nostra Costituzione lo stato di emergenza non è previsto. Lei si è prodigato durante il suo discorso a giustificare lo stato di emergenza, perché altrimenti decadrebbero determinati provvedimenti piuttosto che altri, ma in realtà dovrebbe ammettere ci sono stati altri periodi duri nella Repubblica italiana e che qualcun altro, a differenza sua, ha utilizzato gli strumenti giuridici attualmente in essere per far fronte a quelle emergenze.

«La nostra Costituzione non contempla un diritto speciale per lo stato di emergenza (...) Nella Carta costituzionale non si rinvengono clausole di sospensione dei diritti fondamentali da attivarsi nei tempi eccezionali né previsioni che in tempi di crisi consentano alterazioni nell'assetto dei «La Repubblica ha attraversato varie situazioni di emergenza e di crisi (...) che sono state affrontate senza mai sospendere l'ordine costituzionale, ma ravvisando al suo interno gli strumenti idonei a modulare i principi costituzionali in base alle specifiche contingenze: necessità, proporzionalità, bilanciamento, giustiziabilità e temporaneità Allora, presidente Conte, io faccio un esercizio più per me stessa che non per lei, perché sicuramente lei sa e conosce bene quali sono i diritti costituzionali che ha violato, a cominciare dalla libertà circolazione, alla libertà di riunione, il diritto di professare la propria fede religiosa nei luoghi di culto, il diritto allo studio, la libertà di iniziativa economica, la libertà di espressione di pensiero e, soprattutto, la libertà personale. Presidente, lei ha promulgato lo stato d'emergenza il 31 gennaio e allora io mi chiedo perché il giorno dopo non avete approvato anche un piano pandemico *(Applausi)* da mandare alle Regioni?

avere alcun tipo di piano, alcun tipo di indicazione seria da dare alle nostre Regioni? Ora venite qui e ci chiedete una proroga di ulteriori tre mesi, ora che le cose sembrano andare un pochino meglio. E allora che cosa è che non ci state dicendo per giustificare questa proroga?

non avete sbagliato - come lei dice - quali sono le ragioni che giustificano la richiesta di proroga? O avete informazioni gravi, non state esplicitando a questo Parlamento, oppure avete altri scopi, magari per giustificare o attenuare la partecipazione ad una campagna elettorale che forse magari vi potrebbe mettere un po' in difficoltà. A volte a pensar male ci si azzecca. Allora, dopo sei mesi dal 31 gennaio, noi come Lega abbiamo chiesto al ministro Speranza la settimana scorsa se c'era un piano un piano pandemico; oggi lo avete o pensate di scaricare sui governatori ogni tipo di responsabilità, come è uso di questo Governo? l'obiettivo è dire che la sanità regionale non funziona, ricentralizziamo; buttiamo all'aria una riforma durata quaranta perché dobbiamo ricentralizzare tutto. Noi non ci stiamo però, Presidente. Noi le stiamo chiedendo se avete un piano per gestire l'epidemia *(Applausi)*, per gestire i micro focolai, come se fossero delle microzone rosse. State preparando una campagna di informazione? Sinceramente non si vede nulla. voi dovete queste risposte non solo al Parlamento, ma a tutti gli italiani. Le Regioni ci dicono che hanno il materiale sufficiente per l'ordinario e non per affrontare eventualmente una seconda ondata.

nostro avvocato del popolo, non basta l'apparenza, ma serve anche la sostanza e giace qui un'interrogazione della Lega che chiede quali siano le vostre posizioni rispetto alla tutela dei confini, sia aerei che terrestri terrestri e marittimi. Il ministro Speranza ha firmato l'ordinanza. Apprendiamo quotidianamente che ci sono diversi focolai ovunque - come ha detto anche lei - in Baviera, in Bosnia, in Croazia, in Polonia e Romania.

avevate sottoscritto un accordo con Malta, facendo quello che l'ex ministro Salvini non aveva fatto e ottenendo la rotazione dei porti, la ripartizione dei migranti e le sanzioni per coloro che non si prendevano i migranti. Ci dite dov'è quell'accordo?

il suo entusiasmo sul *recovery* *fund* non sia un *bluff,* anche se qualche dubbio mi viene perché si sta già ricominciando a parlare di MES. Presidente abbia più a cuore la salute degli italiani. Impedite agli stranieri di fuggire dai centri di accoglienza; abbiate a cuore la salute degli italiani. Girano malati di Covid e voi dovete mettere in sicurezza i nostri concittadini e voi dovete mettere in sicurezza i nostri concittadini e la nostra fragile economia. Non potete nascondervi dietro lo stato di emergenza per limitare le libertà costituzionali. Presidente Conte, gli italiani voteranno e il suo Governo, nato nelle stanze dei palazzi, andrà a casa. E quel giorno voi inizierete a pagare tutti i danni che avete causato.

sul nostro Paese nessuno era preparato: eravamo inermi di fronte al mostro e tutti abbiamo fatto la nostra parte. Gli italiani hanno dimostrato di essere all'altezza della sfida e poter contenere questo nemico invisibile adottando tutte le precauzioni del caso: mascherine, distanziamento e uso continuo dei disinfettanti. Abbiamo conosciuto questo *virus*, lo abbiamo studiato, l'abbiamo osservato e, purtroppo, lo abbiamo anche subito. Abbiamo imparato sintomi, segni e parole a molti di noi sconosciuti; qualcuno ha scoperto il saturimetro, la dispnea e la CPAP. Oggi però la situazione non è quella di qualche mese fa

Cosa c'è oggi di imprevedibile se siamo perfettamente in grado di tracciare contagi e curarli, conosciamo la malattia, abbiamo numerosi letti di terapia intensiva costruiti *ad hoc* e inutilizzati e da mesi conosciamo anche le probabilità statistiche della cosiddetta ondata di ritorno? ritorno? Io non sarò mai una negazionista; non dirò mai che le mascherine non servono più, anche per la mia vita precedente. Anzi, Anzi, sono stata la prima a chiamare imbecilli, forse sbagliando, quei ragazzi che, finito il *lockdown*, si sono buttati in strada mettendo a rischio le vite altrui, con ancora - purtroppo - i nostri cari da piangere. Il Governo però guarda la pagliuzza e non la trave, perché manda gente in tuta mimetica sulle spiagge per controllare le coppie che prendono il sole, mentre nel frattempo centinaia di migranti, di cui molti Covid positivi, scappano dai CARA, per non parlare dei continui sbarchi sulla povera Lampedusa ormai stremata.

Ascolti questa frase: «C'è un evidente correlazione tra immigrazione e Covid. È semplicemente irragionevole ritenere che tutto questo non abbia alcun rapporto con i flussi migratori». Chi lo ha detto? Non certo un esponente delle opposizioni, non certo un pericoloso reazionario, ma l'ha detto il vostro Marco Minniti, il vostro tanto amato ministro dell'interno Marco Minniti, esponente del Partito Democratico. Se non ascoltate le opposizioni, se non ascoltate noi, almeno ascoltate qualcuno che avete già in casa. Forza Italia si è mobilitata a tutti i livelli. Oggi torniamo qui a chiedere al Governo di ripristinare la legalità e di controllare le frontiere - lo abbiamo già chiesto alla Commissione europea) oggi il virus viaggia attraverso il Mediterraneo sui barconi *killer*, che continuano a sbarcare, ma anche lungo la cosiddetta rotta balcanica e sui voli provenienti da Paesi particolarmente a rischio. Se non si interverrà, finiremo travolti. Signor Presidente, a febbraio voi eravate tutti giustificati, perché - come ho detto in precedenza - non si sapeva; ma d'ora in poi non lo sarete più. Sia chiaro: il livello di guardia deve rimanere alto, perché la pandemia non è vinta - lo ripetiamo - ma è sotto controllo. Altro però è diffondere il panico e far sentire gli italiani stretti in una morsa, senza dare alcuna prospettiva certa. Gli italiani vanno incoraggiati e protetti, guidati in questa fase del tutto nuova, ma non impauriti inutilmente. Ecco, forse più che stato di emergenza, gli italiani avevano bisogno di uno Stato di emergenza (con la S maiuscola), di uno Stato, cioè, in grado di sostenere chi si è trovato in difficoltà a causa della pandemia: famiglie, commercianti, liberi professionisti, dipendenti di aziende che sono ormai tecnicamente fallite a causa del *lockdown*. Secondo l'Istat andranno persi più di 3 milioni e mezzo di posti di lavoro; l'economia rischia il collasso; i consumi sono già crollati e protrarre ancora questa contrazione, oltretutto facendo del terrorismo psicologico - perché si chiama così, presidente Conte, checché ne dica lei - rischia di innescare un circolo vizioso dal quale sarà difficile uscire. E non pensate di rispondere a questa situazione drammatica - come ha fatto qualcuno del vostro Esecutivo - dicendo ai ristoratori che possono anche cambiare mestiere, perché noi francamente, e gli italiani pure, siamo stanchi del vostro pressapochismo. C'è anche un secondo aspetto fondamentale da considerare: perché siamo sempre così masochisti da dare all'estero un'immagine del nostro Paese che lo presenta come un potenziale lazzaretto? Come pensate possa rialzarsi e rilanciarsi l'Italia? Questo si traduce in un colpo fatale per le esportazioni, per il *made in Italy* e per i settori vitali del PIL italiano, a partire da quello turistico, che avete già completamente abbandonato in questa pandemia. La paura, forse, è piuttosto che sia proprio il Governo a farsi trovare nuovamente impreparato in caso di una seconda ondata. Avete previsto abbastanza mascherine, test, reagenti e personale in numero sufficiente, vista l'esperienza passata? Parafrasando Brecht, beato il popolo che ha bisogno non di eroi, ma di infermieri e medici ben pagati, quelli sì. *(Applausi)*. E veniamo a un altro grande fallimento del Governo, l'*app* Immuni. Rilasciata in grave ritardo, non ha raggiunto il *target* e quindi risulta inutile, nonostante tutta la potenza di fuoco comunicativa. È stata scaricata da 4,4 milioni di persone;

avvertirne 23. Complimenti! Nel novero di quelle che si stanno rivelando delle armi a doppio taglio e per cui lo stato di emergenza sarebbe un'ulteriore mazzata, c'è il prolungamento dello *smart working*, che si sta trasformando in una vera e propria forma di costrizione tra le mura domestiche. Le donne si sono trovate a svolgere in contemporanea ruoli di madri, lavoratrici, insegnanti, a fronte di un tempo di lavoro che si è dilatato fino alle ore notturne per garantire la stessa la stessa redditività; un effetto perverso, considerata anche la perdita di 250 milioni al mese da parte del nostro sistema economico e commerciale. Da Presidente della Commissione infanzia, non posso che invitarvi a una riflessione sui bambini. Questo *lockdown* ha privato bambini e adolescenti di quelle abitudini che costituivano la loro vita quotidiana; il senso della perdita costante li ha resi molto vulnerabili.

per continuare con i vostri fallimenti, non possiamo dimenticare le continue incertezze sulla scuola Non siamo macronisti e nessuno può certo dire che Macron sia il nostro faro, ma gli riconosciamo di essersi preso la responsabilità politica di aver deciso di riaprire le scuole: ha deciso lui e non ha scaricato la responsabilità su Regioni, prèsidi o *task force*.

per sintomi di Covid, perché a ottobre sarà pieno di bambini con la febbre. Avete previsto l'immunizzazione obbligatoria contro l'influenza per gli studenti, in vista di una possibile seconda ondata? Oppure l'Azzolina non fa che proporre idee completamente inutili, un deserto di soluzioni in cui si arenano le ruote dei banchi innovativi

Diciamo la verità e diciamola agli italiani: la dichiarazione dello stato d'emergenza che oggi chiedete al Parlamento non è per l'interesse nazionale né per la pandemia, ma è semplicemente una questione politica, che serve a voi per continuare a manovrare col favore delle tenebre, che ai cittadini non darà però alcun beneficio. La prova sapete qual è? È sotto sotto gli occhi di tutti: in questi mesi di stato d'emergenza non avete dato un esempio di buon Governo. Tanta è la preoccupazione per questa pandemia, addirittura da chiedere lo stato d'emergenza, che - guarda caso - vi fa affrettare a modificare la legge elettorale in piena estate, anche a costo di dividere la vostra stessa maggioranza

stato d'emergenza. Provate a blindare i vostri posti a scapito della ripresa economica e lo fate sulle spalle di tanti artigiani, commercianti, professionisti e cassaintegrati che non sanno come andare avanti. Diciamolo agli italiani: la settimana scorsa avete rimandato addirittura il voto sul terzo scostamento di bilancio, perché non vi eravate messi d'accordo sulle Presidenze delle Commissioni *(Applausi).* È questa l'emergenza che volete? O volete accentrare e sottrarre l'autonomia ai centri decisionali? Avete levato gli scudi contro Orbán, ma le do un'altra notizia: in Ungheria lo stato d'emergenza è stato già chiuso dal 16 giugno. avvio a concludere: fin dall'inizio di quest'emergenza, ci avete chiesto responsabilità. Siamo responsabili e continueremo ad esserlo. Quindi, non temete, ma - meglio - non devono temere gli italiani: qualora la situazione sanitaria dovesse imporre una nuova necessità, sosterremo senza problemi un nuovo stato d'emergenza, che, per chi non fosse avvezzo alle regole, sarebbe dichiarato in pochissime ore; ma non lo faremo, se ciò non sarà necessario, perché non ammazzeremo l'Italia per farvi sopravvivere sulle vostre poltrone. Presidente, mi permetta un consiglio non richiesto: impari un po' dalla sobrietà del ministro Roberto Speranza, che ha lavorato lontano dai riflettori e dato il suo contributo senza fare lo *show*. Guardi: non c'è partito più lontano dal mio di quello dell'onorevole Speranza e, quindi, non glielo dico

Cassese, che non ha bisogno di presentazioni, dice che questo stato d'emergenza è politicamente annoverabile tra i provvedimenti illegittimi e inopportuni. Signor Presidente, l'ho ascoltata prima: o il professor Cassese ha preso un abbaglio o forse le cose non stanno come le ha descritte lei.

vorrei non dover ricordare a quest'Assemblea cos'abbia significato l'emergenza Covid per l'Italia, ma purtroppo credo sia necessario, perché molti sembrano averlo già dimenticato. sembra averlo dimenticato soprattutto chi intorno alla proroga dello stato d'emergenza ha montato una diatriba politica, cercando di confondere stato d'emergenza con nuovo *lockdown*, per fomentare le paure legittime dei cittadini. Questa pandemia, dovuta alla diffusione di un virus altamente contagioso, ha richiesto un intervento deciso della politica per salvaguardare la sicurezza degli italiani. Eppure, spesso in questi mesi, nonostante il dibattito sulla salute dei cittadini dovrebbe sempre fondarsi su punti di vista analitici e seguire il metodo scientifico, è diventato e continua ad essere oggetto di contrapposizione politica. Oggi, a sei mesi dall'arrivo di questo nemico invisibile e sconosciuto, abbiamo quelle che in scienza chiamiamo «evidenze» e che sopravvengono alle deduzioni iniziali. Abbiamo cioè i dati empirici dell'intera curva epidemiologica per poter tracciare un quadro più chiaro, che non risponde a sentimenti di ottimismo o pessimismo, di sparizione o comparsa del virus, ma che si delinea dai numeri dei contagi, dei ricoveri, dei decessi e dei guariti. Il comportamento di qualsiasi virus, e quindi anche del SARS-Cov-2, è infatti delineato da evidenze scientifiche e di questo virus certamente oggi sappiamo ancora troppo poco, soprattutto riguardo allo sviluppo dell'immunità e agli effetti a lungo termine per chi lo ha contratto. In questi mesi mi sono chiesta spesso quale fosse la responsabilità di un Governo e di un Parlamento in una tragedia simile. E di certo la responsabilità non è essere incautamente ed infondatamente ottimisti, bensì agire con cautela seguendo le indicazioni di medici e scienziati, che continuano a raccogliere evidenze per tracciare il percorso futuro più efficace a tutela della salute pubblica. A marzo, abbiamo visto che, quando la curva epidemiologica saliva vertiginosamente, non avevamo tempo per mettere in pratica tutte le misure consone a fermare i contagi, ed abbiamo imparato che è assolutamente necessaria la tempestività. Oggi tutta l'Europa e il mondo intero hanno riconosciuto nel modello Italia della gestione dell'emergenza una eccellenza da prendere ad esempio al punto che il premio Nobel Paul Krugman, con un editoriale sul «New York Times», ha elogiato il nostro Paese per come ha affrontato l'epidemia da Covid. E noi la ringraziamo, signor Presidente del Consiglio, per essere stato l'uomo giusto al posto giusto. Se avessimo ascoltato chi, a fine febbraio, chiedeva di riaprire tutto, forse oggi avremmo ancora centinaia di morti ogni giorno. Grazie alla competenza e alla dedizione di questo Governo, siamo riusciti ad arrestare i contagi in un paio di mesi, nonostante siamo stati i primi nel mondo occidentale ad essere investiti dalla pandemia e ad oggi contiamo più di 246.000 casi e più di 35.000 decessi. A distanza di tempo, tutte le misure messe in campo, a partire proprio dalla dichiarazione tempestiva dello stato di emergenza, si sono rivelate le più idonee a far calare la curva dei contagi. Ce l'abbiamo fatta perché, nonostante politiche decennali di tagli operati nel settore della sanità, abbiamo potuto contare sulle nostre risorse umane, le nostre eccellenze, il nostro personale sanitario, che ha agito compatto con il giuramento di Ippocrate stampato a fuoco sul cuore e ha operato instancabilmente giorno e notte con spirito di sacrificio immolandosi: non posso usare altro termine visto l'ingente numero di vite umane che abbiamo perso tra le fila di coloro che per mesi abbiamo chiamato «eroi». Ce l'abbiamo fatta perché, nonostante l'indole libera ed indomita che ci portiamo scritta nel codice genetico, abbiamo osservato le regole; siamo stati rispettosi e diligenti; abbiamo riscoperto un sentimento di coesione e ritrovato la bellezza della solidarietà che antepone il noi all'io. Ce l'abbiamo fatta perché gli italiani ci hanno dato fiducia nonostante le sofferenze e le grandi difficoltà; hanno creduto in lei, signor Presidente del E noi ci siamo messi all'opera da subito senza mai fermarci, e non solo per tutelare la salute e arginare l'epidemia, ma anche per fronteggiare i danni economici e sociali derivanti dalla pandemia. Ce l'abbiamo fatta sicuramente perché l'uso delle mascherine e le misure di distanziamento sono stati strumenti efficacissimi per ridurre la carica virale in circolo e permettere la riapertura graduale in sicurezza, evitando una nuova immobilità. I numerosi focolai diffusi sul territorio nazionale ci chiedono, però, di mantenere alta la guardia e di rispettare l'indicazione di indossare le mascherine nei luoghi chiusi e affollati. Eppure, c'è chi lamenta che anche questo sia troppo. Presidente, io queste persone le porterei nei reparti di terapia intensiva nel momento di massimo affollamento *(Applausi)*, con i pazienti attaccati ai respiratori, completamente nudi in posizione prona, soli, lontani dai propri cari per settimane e, a volte, per sempre. sempre. Sono certa che chi ha vissuto questo errore e questo dolore non può dimenticarlo e di certo non lo dimenticano gli occhi dei nostri operatori sanitari, che ci chiedono di rispettare il loro impegno e il loro sacrificio, non con la propaganda o con le promesse, ma con il nostro buon esempio, soprattutto nelle sedi istituzionali. Opporsi alla proroga dello stato di emergenza può solo essere un atto politico, Presidente, e non una scelta razionale, perché stato di emergenza significa dare la possibilità al Governo di prendere decisioni in modo tempestivo. Eppure, abbiamo sentito dire in quest'Aula che non serve. A chi non serve? Non serve ai malati? Non serve agli operatori sanitari, ai commercianti, che non vogliono dover abbassare di nuovo le serrande, alle imprese? O non serve a cittadini della Lombardia, che hanno visto morire più di 16.000 persone e oggi devono assistere ad indagini su tentate speculazioni nella gestione di questa emergenza? *(Applausi)*. Signor Presidente, io dico che serve. Serve certamente ai cittadini italiani sapere che, se dovesse essere alto il rischio di compromissione della salute pubblica, allora il Governo potrà agire con tempestività, perché la tempestività è stata la nostra salvezza. Non possiamo permetterci un nuovo sovraccarico del nostro Servizio sanitario nazionale, prima di averlo potenziato; un altro sacrificio dei nostri medici, degli infermieri, dei volontari; non possiamo permetterci un nuovo *lockdown*. E mi auguro che che questo sia il pensiero condiviso da tutti, perché per tutelare il bene dell'Italia e degli italiani nella scienza e nella medicina bisogna agire razionalmente. E, se non sappiamo ancora bene come curare questo virus, certamente sappiamo di avere un Governo responsabile e un Servizio sanitario nazionale reso più forte proprio da questo Esecutivo. Sono questi i due pilastri su cui costruire la nostra sicurezza e porre le basi per la ripresa di un'Italia che adesso ha davvero bisogno di splendere. *(Applausi)*.

Faraone e Unterberger, e n. 2, dai senatori Romeo, Bernini e Ciriani. I testi sono in distribuzione. Avverto che è in corso la diretta televisiva con la Rai.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 Signor Presidente, gentili senatrici e gentili senatori,

e delle varie argomentazioni, preferendo poi intrattenermi per ascoltare con molta attenzione tutti gli interventi. In questo caso ne approfitto e faccio un'eccezione. Ho ascoltato alcuni interventi, in particolare dell'opposizione, colorati di venature polemiche, direi finanche ideologiche, su un tema in discussione che mi ero permesso di classificare anche come una questione

Certo, questo non deve essere un dibattito tra cultori del diritto costituzionale; ci sono dei pro e dei contro ed è una delle ragioni per cui abbiamo dovuto costruire un percorso normativo *ad hoc* *ad hoc* che non era previsto in particolare nel dettato costituzionale. Non dobbiamo, però, confondere il fatto che non ci sia un percorso *ad hoc* nella nostra Costruzione con il fatto che non si debba intervenire per adottare misure e perseguire un *iter* normativo specifico nel segno evidente della tempestività e dell'efficacia degli interventi normativi e anche operativi. Quando si dice che nella Costituzione non è previsto lo stato di emergenza, non si può concludere che sia illegittima la proclamazione dello stato di emergenza. Invito di nuovo a considerare che forse non ce ne siamo accorti, ma dal 2014 ad oggi abbiamo dichiarato lo stato di emergenza 154 volte, e lo abbiamo prorogato per 84 volte. Quindi, lo stato d'emergenza è previsto da una norma di rango primario nel decreto legislativo n. 1 del 2018, il nostro codice della Protezione civile. Allora non deve apparire un fuor d'opera il fatto che si imponga la necessità di prorogare uno stato di emergenza dichiarato ai sensi del codice della Protezione civile. Se lo proroghiamo infatti eventi verificatisi molto lontano nel tempo e fatti specifici isolati come possono essere un'alluvione o un terremoto, ancor di più, forse, è giustificata una proroga per un evento come la pandemia che - e siamo tutti d'accordo in questo momento - stiamo contenendo, perché la curva epidemiologica è assolutamente sotto controllo, e ci auguriamo che rimanga sotto controllo. La pandemia, però, è pur sempre un evento che si sviluppa in modo continuo e imprevedibile perché il virus continua a circolare. circolare. Ho chiarito - a qualcuno però sfugge e continuo quindi a ripeterlo - che stiamo ragionando perché la dichiarazione dello stato di emergenza ci consente di attivare nel nostro ordinamento giuridico una serie di misure organizzative, operative e funzionali che ci permettono di garantire piena assistenza e protezione a tanti soggetti attualmente esposti in modo diretto e indiretto agli effetti della pandemia. In particolare, ho cercato di sottolineare - evidentemente non sono stato chiaro e quindi preferisco precisarlo che tra le misure organizzative, operative e funzionali ci sono interventi che riguardano direttamente il capo della Protezione civile e il commissario straordinario che in questo momento ci consentono di completare il progetto di potenziamento delle strutture ospedaliere, che francamente lasciare a metà dell'opera sarebbe assolutamente sconveniente e controindicato. Ci consentono di perseguire il piano di sicurezza delle nostre scuole, perché immagino che tutti vogliamo che i nostri studenti, i nostri ragazzi e ragazze possano tornare a settembre a scuola in piena sicurezza. Ci consentono finanche - è cronaca delle ultime ore che anche le forze di opposizione siano particolarmente sensibili al tema - di perseguire con tempestività ed efficacia un piano di sorveglianza sanitaria dei migranti. alla luce delle norme attuali, abbiamo addirittura difficoltà ad operare una requisizione di navi traghetto dove vorremmo ovviamente assicurare lo svolgimento delle quarantene e, quindi, programmare un'adeguata ed efficace

Ho parlato, quindi, di una proroga dello stato di emergenza imposta da ragioni squisitamente tecniche, ma non volevo intendere - come qualcuno dell'opposizione ha sottolineato - che volevo precludere una valutazione politica. Ci mancherebbe!

e anche ovviamente il pieno ripristino e la più sicura ripartenza di tutte le attività economiche, sociali e culturali. Attenzione: noi oggi ci avviamo a questo perché abbiamo tutto un sistema di protezione; molte delle misure non sono visibili, ma io vi sfido vi sfido anche a interrogare gli stessi Presidenti di Regione, che sono soggetti attuatori per quanto riguarda dette misure rispetto al capo della Protezione civile;

dovrebbe imputare al Governo la volontà di prorogare lo stato di emergenza per alimentare paure, allarmismi - come pure purtroppo ho sentito - o ancora addirittura per la velleità di provocare torsioni autoritative del nostro sistema democratico. Credo che si possa essere in disaccordo con le azioni del Governo, con le attività e le iniziative assunte, ma ci darete atto che sin dall'inizio della pandemia questo Governo ha agito in piena trasparenza; è venuto sempre in quest'Aula a confrontarsi con il Parlamento; ha definito un percorso garantista

Dal 18 maggio, quando questo Governo si è assunto la responsabilità di allentare le misure restrittive e di consentire la piena riapertura di tutte le attività, on ci avete più sentito parlare di allarme sociale, di pericoli vari, eccetera. Noi stessi abbiamo creato e stiamo mantenendo quelle misure minimali di precauzione, come la regola sul distanziamento, che adesso ci consentono di correre. L'Italia deve correre.

da condividere, a prescindere dalla maggioranza e dall'opposizione. Mi avvio pertanto alla conclusione dicendo che abbiamo seguito un metodo dall'inizio. Se ci viene riconosciuto anche all'estero di avere superato con una certa efficacia il periodo più acuto della crisi, è perché questo Governo dall'inizio ha seguito un metodo. Ha seguito il metodo del principio di precauzione, della trasparenza con tutti, Parlamento e cittadini, il principio dell'adeguatezza e della proporzionalità delle misure adoperate. Abbiamo cercato di non adottare misure sovradimensionate e soverchie e di adottarle quando davvero si palesavano come necessarie per ottenere lo scopo di contenimento del contagio. Adesso vi invitiamo a considerare la necessità di prorogare lo stato di emergenza, ancora una volta senza nessun allarmismo, senza nessuna volontà di alimentare paure, ma semplicemente per l'opportunità, anzi, la necessità di continuare a mantenere questo apparato di misure minimali che ci consentono di correre e, in particolare, di conservare piena efficacia e tempestività di intervento a questo apparato. Ripeto che la valutazione è di ciascun singolo parlamentare, in piena coscienza e in piena assunzione di responsabilità. Per quanto riguarda le risoluzioni

(SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, nella situazione eccezionale che stiamo vivendo, io credo che un solo principio debba guidare le scelte del decisore pubblico e questo principio si chiama buon senso. purtroppo, noi assistiamo ad un dibattito che lascia veramente molto perplessi. Scorrendo i giornali e il *web* in queste settimane non sono pochi quelli che dicono che il virus è passato, compiendo una drammatica opera di rimozione di quanto accaduto. Allora, conviene partire da quello che sappiamo, anzi, da quello che non abbiamo: non abbiamo dati coerenti sulla gestione del virus. Dal punto di vista terapeutico ci sono ancora molti dubbi. Non è chiara la risposta immunologica all'infezione. Quindi, anche la valenza dei test immunologici è ancora molto dubbia. Non abbiamo, soprattutto, il vaccino, con un percorso ancora impegnativo in questo senso, anche se negli ultimi giorni i dati scientifici fanno ben sperare. Quindi, fino al giorno in cui ci sarà, finalmente, il vaccino, tutti noi dovremo convivere ancora con questo virus. È più semplice per quei Paesi, come l'Italia, che hanno buoni dati sulla diminuzione dei contagi; più complicato per quelli che vedono drammaticamente aumentare il numero dei malati e dei morti. C'è un filo rosso che lega tutti i Paesi come gli Stati Uniti, il Brasile e il Regno Unito, dove la curva dei contagi è ancora alta,

non dobbiamo cadere nella stessa tentazione; e anch'io voglio ricordare con piacere il bellissimo *reportage* del «New York Times»: l'Italia da malato d'Europa ha dimostrato al mondo come si può guarire e questo grazie all'azione lungimirante del suo Governo. Questo è merito, appunto, del principio prudenziale che ha mosso il Governo, che ha dichiarato lo stato d'emergenza quando nel nostro Paese c'erano due soli casi - ricordiamo la coppia di cinesi ricoverati allo Spallanzani e mancavano ancora tre settimane alla scoperta di primi focolai in Lombardia e in Veneto. Mi chiedo allora perché, oggi che siamo di fronte a centinaia di casi al giorno, con un quadro internazionale decisamente peggiore di quello dello scorso gennaio, si debba rendere più lenta e farraginosa tutta la macchina, non prorogando lo stato di emergenza. La proroga di questo stato d'emergenza consentirebbe, appunto, di completare la riorganizzazione del sistema sanitario nel territorio, dalle RSA alla telemedicina, alle strutture ospedaliere dedicate, nell'ottica di un adeguamento rispetto ai vari scenari dell'autunno. Inoltre è l'unico modo per mettere in sicurezza gli ambienti scolastici e garantire un'ordinata apertura dell'anno scolastico. Bambini e adolescenti mancano da quei banchi da più di duecento giorni ed è qualcosa di inaccettabile, se pensiamo che il 13 per cento di loro non ha avuto la possibilità di accedere alla didattica a distanza. Attraverso lo stato di emergenza si possono tenere in vita tutte le disposizioni volte a garantire il distanziamento sociale, a cominciare dall'utilizzo di dispositivi individuali di protezione. Non nascondiamoci dietro ad un dito: da questo punto di vista, soprattutto in alcuni contesti, oggi si fa una gran fatica a farle rispettare e sarebbe ancor peggio se dicessimo che tutto questo non è più un obbligo, ma una facoltà dei singoli. Per concludere, signor Presidente, sono considerazioni di questo tipo che dovrebbero muovere il pensiero pubblico, cui aggiungo una quarta considerazione: l'impegno per reprimere sul nascere un'eventuale seconda ondata è di vitale importanza, per non vedere la crisi economica tramutarsi in una depressione economica e sociale. sociale. In poche parole, occorre cercare di evitare un secondo *lockdown* in autunno. Il tutto va fatto dando anche maggior fiducia ai territori: le autonomie locali e le Regioni a Statuto speciale, che qui noi rappresentiamo, infatti essere determinanti, potendo esercitare le loro competenze nel gestire al meglio le esigenze di tutti cittadini. Vogliamo quindi ribadire il pieno rispetto dei nostri Statuti di autonomia. Concludo, signor Presidente, citando la metafora che usa spesso il ministro Speranza, che secondo è me di grande pertinenza: l'Italia è come una nave che ha abbandonato la tempesta, ma che non è ancora approdata in un porto sicuro. significa dire ai più forti, ai più giovani e a tutti coloro che godono di buona salute e che troppo spesso tendono a evitare l'obbligo di proteggersi, che il raggiungimento di quel porto sicuro vuol dire stare dalla parte degli anziani, dei disabili, degli ammalati cronici, dei bambini e di tutti coloro che sono particolarmente vulnerabili. Il nostro comportamento responsabile è rivolto a loro e alla memoria delle 35.000 persone, che ci hanno lasciato. Per tutte queste ragioni, signor Presidente, il Gruppo Per le Autonomie sosterrà il Governo sulla richiesta di proroga dello stato di emergenza.

ma mi consentirà di dire che è strano che lei replichi in televisione a qualcosa che i telespettatori non hanno potuto ascoltare. È veramente una caratteristica tipica della sua personalità, ammirevole per tanti versi. che il prolungamento dello stato di emergenza sia indispensabile e necessario, perché altrimenti verrebbero meno l'assistenza e la protezione, non potrebbe completare la protezione civile e il piano di sicurezza per la scuola e non potrebbe bloccare i migranti, che non si sa quando mai li ha bloccati, visto che continuano a scappare, senza che facciate assolutamente nulla. *(Applausi)*. E non ne ho sentito parlare in nessuno degli interventi della sua maggioranza: se la sono presa con i ragazzi che fanno gli aperitivi e con i tifosi del Napoli, ma guai a parlare delle delle fughe dei migranti! Ma questo non importa. Si è parlato poi delle carceri e della sicurezza: ma davvero lei ritiene che per fare queste cose ci sia bisogno di uno stato di emergenza? Lei è laureato in giurisprudenza, addirittura è l'avvocato del popolo e sa benissimo che la nostra Costituzione, nei casi di urgenza, che non hanno niente a che vedere con l'emergenza, prevede il decreto-legge, che lei può attuare immediatamente e che solo successivamente il Parlamento può decidere se ratificare, convalidare, confermare Quindi non ci venga a dire cose che lei sa non essere vere. In altri termini, potrei anche dire - se non apparissi offensivo - che lei mente sapendo di mentire. mentire. Vede, Presidente, noi non abbiamo la minima pretesa di dire che il coronavirus sia completamente debellato; non abbiamo nessuna pretesa di consigliare agli italiani di evitare le precauzioni normali, quelle del buon senso. Ma nello stesso tempo non accettiamo che siano impauriti, che siano messi all'angolo, che siano imbavagliati su presupposti inesistenti. Lei sa molto meglio di me che non ci sono più, da giorni, decessi, neanche per malattie antiche; lei sa benissimo che da due mesi non ci sono casi sintomatici; lei sa benissimo che in questo momento il ceppo dominante del virus è tale da non creare nessun pericolo clinico; lo sa benissimo perché lo dicono le emergenze scientifiche. Certo, poi ci sono i bollettini terroristici, che non possono fare a meno di dire «zero decessi», ma sommano casi sintomatici con asintomatici, casi pregressi con casi attuali; purtuttavia, purtuttavia, emerge chiarissimo che in questo momento lei può solo parlare di un pericolo futuro - certo, ci può essere - di ripresa del virus. Ma lei sa benissimo che uno stato di emergenza - non c'è bisogno che ce lo insegni il professor Cassese è valido solo quando è attuale. Non si può immaginare uno stato di emergenza per un pericolo che verrà, altrimenti, cari colleghi, come qualcuno ha detto, lei ha parlato dei morti, dei feriti, delle sofferenze che tutti abbiamo subito (mica solo la maggioranza) e che tutti abbiamo condiviso (e lei per primo sa che le abbiamo approvato anche gli scostamenti del bilancio), ma non è che, nel ricordo delle sofferenze, possiamo immaginare che per sempre ci sia uno stato di emergenza, quando non c'è più. Significa tenere sotto scacco, sotto paura gli italiani. Ma non era la destra quella che soffiava sul fuoco, quella che giocava con la paura? Avete imparato una lezione che noi non vi abbiamo mai dato. Continuate a giocare con la paura, non vi dico a soffiare sul fuoco, ma è gravissimo quello che state ancora facendo. Siamo gli unici

Si ricorda la sinistra di aver addirittura detto che gli avremmo dovuto sospendere gli aiuti europei, perché con una legge - quella sì -costituzionale (che noi non abbiamo nella nostra Costituzione) si era preso poteri minori di quelli che si è arrogati questo Governo e che gli abbiamo consentito, nel momento di vero pericolo? Ebbene, Orbán e l'Ungheria hanno cessato, con un voto parlamentare, lo stato di emergenza noi lo proroghiamo? Forse non ci importa che questo comporti un rischio per l'Italia di apparire l'untore dell'Europa? Non ci importa che questo provochi un danno economico notevole? Lei infatti sta dicendo al mondo che in Italia c'è uno stato di emergenza che non esiste più, in questa veste; non è che non il pericolo di futuri contagi o l'obbligo di stare attenti, ma non esiste una condizione attuale che giustifichi l'allarme che voi create con questo stato di emergenza. Io potrei proseguire, elencando i numeri e le irregolarità che sono state fatte, la doppia verità di chi era troppo aperto, quando bisognava chiudere (ve lo ricordate all'inizio? Ve li ricordate, cari amici del PD, gli aperitivi sui Navigli, a Milano?), e che adesso, che invece bisogna riaprire, vuole chiudere! *(Applausi)*. Sorge il sospetto che, più che un interesse a mantenere sotto controllo il virus, vi siate inorgogliti dell'aumento di popolarità che ne è derivato. Sapete, quando c'è la paura, anche una bella presenza fisica, un buon eloquio e una rassicurante posizione di certezza aiutano; ma non è che per dare risultati al Governo e alla maggioranza possiamo imbavagliare l'Italia a vita.

proposte su come spendere i soldi che arriveranno, se e quando arriveranno. Siamo pronti a esaminare le necessità figlie di questa terribile evenienza che è alle spalle, e che speriamo non debba tornare; ma se tornasse, saremmo pronti. Ma siamo altrettanto pronti, caro Presidente, a dirle con tutta la nostra chiarezza che abbiamo il sospetto fondato, avvocato Conte, che anziché difendere la causa del popolo italiano, lei stia cercando di difendere la sua popolarità, la sua poltrona e quelle del suo Governo, che non ha la fortuna di avere un voto popolare. Lo cerchi. Se

in maniera chiara, che ci quadra relativamente e che naturalmente i sovranisti non potranno mai dirle.

di prorogare lo stato di emergenza sanitario e non si ritiene di utilizzare le risorse destinate all'emergenza sanitaria che attualmente l'Europa ci mette immediatamente a disposizione. È questa la vera contraddizione su cui dobbiamo dare una risposta, Presidente. Perfino Salvini è coerente nella sua incoerenza: l'uomo che sul coronavirus si è comportato un po' come quel tizio della barzelletta al quale veniva chiesto di affacciarsi dal finestrino

pappalardiana dei gilet arancioni, ci dice che l'emergenza non c'è tranne che per gli immigrati, Presidente: si può girare senza mascherina, non c'è alcun rischio, però tutte le imbarcazioni che arrivano dal Nord Africa sono piene zeppe di contagiati. Salvini un elemento di coerenza ce l'ha: dice che l'emergenza non c'è - nell'attuale deriva pappalardiana - quindi dice coerentemente che non gli servono le risorse economiche del MES, che sono messe a disposizione per il nostro Paese proprio per la gestione di questa fase, Presidente. L'elemento di incoerenza sta qui, di fronte alla disponibilità economica per gestire la fase che lei ha descritto benissimo, e che naturalmente comporta talune necessità di investimento da parte di questo Paese. Tutte le cose che lei ci ha elencato, Presidente, e noi abbiamo la possibilità di utilizzare quelle risorse che servono ora e che dovremmo utilizzare immediatamente, avendo quelle come disponibilità immediata. Quindi, da un lato, si dice che c'è bisogno di uno strumento che consenta di gestire il ritorno eventuale di focolai, l'eventuale chiusura di nuove zone rosse, la possibilità di fare gare, l'avvio dell'anno scolastico, dall'altro lato, niente MES, che è senza alcuna condizionalità. Io credo che questa scelta sia sbagliata e sia puramente ideologica. Sono due comportamenti contraddittori che ci fanno apparire, Presidente, anche meno credibili in Europa. Non è che abbiamo chiesto l'elemosina a qualcuno perché siamo un Paese di pezzenti, noi siamo la terza economia del continente. Se abbiamo chiesto una mano all'Europa, è semplicemente perché il nostro Paese è stato tra i più colpiti dalla pandemia. Solo per questo. Quindi dare la possibilità ai sovranisti o ai frugali di dire che noi abbiamo chiesto una cortesia agli altri Paesi, perché abbiamo una disponibilità,

Anche perché, Presidente, io le ricordo che queste risorse possono essere utilizzate per spese sanitarie, sia dirette che indirette. Per tutte quelle che lei ha elencato, le posso fare anch'io un elenco di spese sanitarie indirette che possono essere sostenute economicamente da quelle risorse. Se pensiamo agli imprenditori, tutto ciò che riguarda la sicurezza delle aziende, sono spese sanitarie indirette. Se noi utilizzassimo quelle risorse per sostenere imprenditori costretti a mettere *plexiglass*, ad allargare i tavoli dei ristoranti per consentire il metro di distanza, per sanificare, se noi dessimo agli imprenditori queste risorse economiche, probabilmente eviteremmo il fenomeno che si sta verificando che vede imprenditori costretti ad aumentare i prezzi, a danno dei consumatori, proprio perché non ce la fanno. Quindi quelle risorse ci servirebbero ora per un interesse diretto degli imprenditori, per favorire una ripartenza. Così come l'avvio dell'anno scolastico. Nello scostamento metteremo risorse che andranno a debito dello Stato destinate all'avvio dell'anno scolastico; anche lì spese indirette per la sanità, risorse che potremmo utilizzare con i fondi del MES. tutto quello che riguarda la riapertura degli uffici pubblici, per chiudere questo terribile *smart working*. Io credo che noi abbiamo l'opportunità di intervenire. riguarda l'anno scolastico, Presidente, continuo a sentire le rassicurazioni del Ministro e mi vanno bene, dopo di che però, girando e ascoltando anche dirigenti scolastici, ne sento tanti che mi dicono che stanno selezionando quali classi fare ripartire. Così come sento tanti genitori che dicono che vanno a iscrivere i loro figli negli istituti scolastici più grandi, dove c'è maggiore possibilità di rispettare le regole. Ciò vuol dire che noi, da questo punto di vista, dovremmo avere una maggiore attenzione e fare un maggiore investimento sulla scuola. Presidente,

Anche lì, quelle sono spese sanitarie indirette e sentire il ministro Lamorgese che dice che non ha la possibilità, perché economicamente non ce la fa, di prendere le navi da crociera

Dio non lo voglia, ma può capitare che noi dovessimo avere bisogno ulteriormente di quell'intervento e tante Regioni del Paese sono impreparate. I medici, il ministro Speranza, gli infermieri; come svuotiamo l'imbuto degli specializzandi? Tutti quei ragazzi che dovrebbero cominciare a lavorare e che sono invece ancora lì che non possono farlo perché non abbiamo le risorse economiche per le scuole specializzazione. Anche per quelli: le risorse del MES.

per cambiare fase bisogna anche cambiare messaggio, perché se noi raccontiamo al Paese che c'è la stessa situazione di quando eravamo in pieno *lockdown* commettiamo un errore. Da questo punto di vista, il linguaggio del suo intervento è stato assolutamente equilibrato.

un passaggio che abbiamo fatto inserire nella proposta di risoluzione per quanto riguarda le strutture residenziali psichiatriche. Continuiamo a ricevere innumerevoli segnalazioni di donne e uomini - mamme e papà che non riescono a ricongiungersi con i ragazzi chiusi e segregati nelle strutture sanitarie psichiatriche, che sono l'ultimo luogo che è rimasto in totale *lockdown*. sono tantissime e noi, presidente Conte, le chiediamo di intervenire affinché anche lì si ritorni alla normalità e si consenta a queste persone di potersi riabbracciare. Mi ha colpito tantissimo la dichiarazione di una mamma che ha detto che suo figlio,

Signor presidente Conte, nel suo intervento ha voluto sgombrare il campo da una serie di interpretazioni,

Gli italiani ci ascoltano ed è giusto che sia chiaro quello che stiamo facendo: la proroga dello stato di emergenza non è il *lockdown*, né gli interventi adottati nei mesi precedenti, che stanno alle nostre spalle. Lo stato di emergenza è un impianto normativo

su un altro impianto normativo che ci faccia uscire da quel linguaggio - stato di emergenza - e ci consenta di disporre delle norme per poter agire. Ma oggi siamo qui

di crescita, sviluppo e riavvio dei lavori nel nostro Paese. Esso non comporta - lo dico ai colleghi - automaticamente nessun intervento normativo che metta dei limiti alla libertà. Come ha detto chiaramente il Presidente del Consiglio e come anche noi, con la maggioranza, ribadiamo nella proposta qualsiasi intervento che si dovesse rendere necessario da questo punto di vista ha bisogno di una fonte normativa primaria, quindi di un decreto-legge, nel rispetto del ruolo del Parlamento e della discussione in Parlamento. Da questo punto di vista, colleghi, non capisco per quale ragione stiamo facendo un dibattito

L'argomentazione poi, tutta politicista, secondo la quale si usa lo stato di emergenza per zittire il dissenso - come è stato detto in questo dibattito dire che è una sciocchezza. D'altra parte l'avete fatta la manifestazione in piazza del Popolo. *(Applausi).* Magari non raggiungendo quel successo che pensavate, ma l'avete fatta; nessuno ve lo vieta e nessuno ve lo vieterà. Non diciamo sciocchezze. Così come è una sciocchezza l'idea secondo la quale lo stato di emergenza è funzionale a puntellare il Governo e senza di esso il Governo cadrebbe. Non è così: la maggioranza c'è la maggioranza c'è ed è solida. Discute a volte in modo non proprio eclatante, non proprio al meglio; potremmo fare meglio, ma la maggioranza c'è. Non esiste, da questo punto di vista... La poltrona? Siamo tutti a sedere su una poltrona, ragazzi, basta con questa demagogia. *(Applausi)*. È demagogia, che non serve agli italiani e all'Italia. Io dico: prima gli italiani e prima l'Italia, prima delle vostre polemiche. *(Applausi)*. Ora, non drammatizziamo ciò che non è. una preghiera a tutti noi. Non voglio fare polemiche, ma evitiamo di fare letture veramente strumentali. L'uso della mascherina è utile e il distanziamento è necessario;

comportamenti che possono creare problemi a tutti noi. E dunque, se ciò è fatto da chi ha responsabilità in questo Paese, è un comportamento - fatemelo dire - irresponsabile e pericoloso. Detto questo, c'è la crisi economica. Questo Paese ha dei problemi e nessuno di noi li nega;

stato fatto da diversi Paesi; e avete visto quali sono i risultati. È stato fatto anche qui in Italia, non solo per gli aperitivi, come è stato citato da qualcuno, ma anche da chi diceva, alla fine di febbraio, di riaprire tutto. Per fortuna che non l'abbiamo fatto! *(Applausi)*. E questo, per onestà intellettuale, dovremmo avere tutti la capacità di riconoscerlo. Ho già detto che dovremmo fare un'analisi sul percorso che ha fatto questo Paese, riconoscendo il valore dei medici e del Sistema sanitario lo sforzo degli italiani. Certo, dovremmo ragionare anche sugli errori e sui limiti. Non c'è dubbio, però, che, per fortuna, gli italiani hanno capito che la scelta fatta dal Governo era giusta. Da questo punto di vista, non preoccupatevi dei dei sondaggi e del consenso del Presidente del Consiglio, perché, se l'esito di questo impegno e lavoro è stato utile per l'Italia, dobbiamo ringraziare il Governo. *(Applausi).* E stimolarlo adesso a uscire dalla logica dell'emergenza e impostare una visione. Il nostro dibattito, colleghi, infine,

proporre per l'Italia, non sulle cose emergenziali, ma su quale visione abbiamo del sistema fiscale, dell'equità fiscale, delle politiche industriali e del cambiamento che deve fare questo Paese? Quale idea abbiamo? Dovremo discutere di questo, perché siamo stati eletti per dare un futuro al Paese, non solo per cavalcare la propaganda o magari avere un qualche *tweet* o consenso in più in un sondaggio.

l'Organizzazione mondiale della sanità dichiara l'emergenza sanitaria; il 31 gennaio, subito dopo, il Governo italiano fa altrettanto: dichiara lo stato d'emergenza e lo fa per sei mesi. Quello di cui discutiamo oggi è se serve prorogare ulteriormente lo stato d'emergenza. Vorrei fare un passo indietro, in modo che tutti in quest'Aula facessimo memoria di quello che abbiamo vissuto in questi mesi,

siamo abituati a darci la mano, quando ci incontriamo, e ad abbracciare le persone che ci sono care. Da un momento all'altro, abbiamo dovuto cambiare la qualità delle nostre relazioni e modificare abitudini consolidate (come imparare a lavarci le mani e sanificare gli ambienti).

ricordato. Vorrei che tutti lo ricordaste, come ricordo il giorno in cui sono entrata in quest'Aula e ho visto tutte le persone con la mascherina: mi sembrava di essere entrata in un film di fantascienza; non potevo credere che stesse succedendo a noi; davvero non lo pensavo possibile ed è stato un momento di straniamento incredibile. Poi tutti in casa, con il *lockdown*: le scuole chiuse; i luoghi di culto chiusi; gli stadi chiusi; al lavoro non si poteva più andare;

Nelle strade in quei giorni si sentivano soltanto le sirene delle ambulanze, molte, incessanti. I nostri operatori sanitari, i cui volti vedevamo vedevamo tumefatti dalle mascherine e dalla stanchezza, stavano reggendo una situazione di estrema difficoltà, perché neanche la sanità era pronta a quella pandemia; in modo molto rapido, però, e con atti di eroismo veramente incredibile, le strutture si sono adattate e hanno messo necessaria revisione dei padiglioni per accogliere le emergenze. Ci sono stati turni defatiganti e impossibili che i nostri operatori, i nostri medici e tutto il personale della sanità hanno fatto; e si sono trovati spesso spesso da soli a dover confortare persone che da un momento all'altro sono uscite dalle loro case, si sono ammalate, sono entrate in un ospedale, non hanno più potuto vedere i loro cari e sono morte. Ripeto, i loro cari non li hanno più visti e l'ultima mano è stata quella di un operatore sanitario che li ha guardati negli occhi andare via. Abbiamo scoperto che i dispositivi di tutela individuale - all'inizio c'era difficoltà a trovare le mascherine e i camici - sono produzioni strategiche come quelle che pensiamo per la Difesa (nella Difesa siamo abituati a immaginare che ci siano alcune produzioni considerate strategiche). Dobbiamo ripensare al fatto che ci sono produzioni che riguardano la sicurezza che sono strategiche. Abbiamo avuto più di 35.000 morti e nessuno può dimenticare quell'immagine incredibile dei camion dell'Esercito che portano via le bare. In quel momento il Paese guardava tutto attonito. Ed io ricordo anche in quest'Aula la vicinanza agli operatori sanitari, ma anche la commozione perché molti di noi hanno avuto amici che sono stati colpiti, si sono ammalati e alcuni purtroppo non ci sono più. Perché ricordo tutto questo? Perché non è qualcosa lontano nel tempo: sono passati appena tre o quattro mesi. Certo, l'emergenza sanitaria fortunatamente si è notevolmente attenuata, perché è stata affrontata con efficacia, ma potrebbe ripartire. Rimettere in moto il Paese, non farlo fermare è un obiettivo di tutti, ma occorrono responsabilità e prudenza. Continuiamo a seguire le regole per la sicurezza di tutti. Anch'io trovo grave che ci siano *leader* politici - ed è avvenuto anche qui in Senato - che danno con i loro atteggiamenti un messaggio assolutamente contraddittorio rispetto a quello che serve. Guardate, lo hanno fatto in altri Paesi, ad Boris Johnson, Trump, Bolsonaro, e non mi pare che abbiano poi dato prove e dimostrazioni; alcuni si sono anche dovuti pentire e lo hanno detto pubblicamente. Quindi evitiamo perché ognuno di noi è un modello per un pezzo di Paese, è seguito; non diamo questi messaggi, perché non è finita. Allora, perché prorogare lo stato di emergenza? È stato detto bene dal Presidente del Consiglio, anche se poi da molti interventi dell'opposizione è stato travisato: è la cornice, il quadro per intervenire con provvedimenti *ad hoc*. È stato spiegato il ruolo delle ordinanze della Protezione civile: sono ordinanze che possono essere fatte immediatamente fuori dai tempi normali solo se c'è lo stato di emergenza. Non è un nuovo *lockdown*; lo hanno detto molti in quest'Aula, ma ricordiamolo: non è la privazione di libertà che è stata necessaria nel momento acuto della crisi. Speriamo di no, ma potrebbero esserci nuovi picchi, e noi dobbiamo con precauzione guardare anche a questo. Comunque, nella transizione dobbiamo mantenere regole comuni e regole prudenti di comportamento, anche perché, come molti hanno ricordato, la situazione internazionale è ancora grave. La fase non è più acuta; giustamente è stato coinvolto il Parlamento e dovrà sempre essere coinvolto: il Partito Democratico è convinto che sia importante questo metodo (questo è il significato della comunicazione di oggi). L'altro elemento è che noi riteniamo che i provvedimenti debbano essere proporzionati all'evoluzione della situazione. Detto tutto ciò, veramente non capisco - non è una questione di posizione di maggioranza - perché si sono alzati i toni, pensando di cavalcare dall'opposizione questo provvedimento come una clava da lanciare nella battaglia politica. Non lo capisco, non lo capisco proprio: sono sincera, non è per oppormi a quello che avete detto. Ma davvero qualcuno pensa seriamente che ci possa essere chi ha interesse a non far ripartire il Paese? Veramente io mi stupisco di voi. Ma potete pensare che prolungare lo stato di emergenza vuol dire ritardare la ripartenza? Non è così. Che qualcuno voglia danneggiare l'immagine dell'Italia? Ma semmai è il contrario: i turisti che vogliono venire in Italia, se vedono un Paese che guarda con attenzione alle regole, è più facile che decidano di venire in Italia anziché andare in un altro Paese dove invece, avendo avuto meno prudenza nelle regole, sono ripartiti purtroppo dei focolai. Oppure davvero, come ho sentito, qualcuno pensa che questo sia un marchingegno diabolico per mantenere il consenso? E perché dovrebbe servire a questo? Il gradimento dell'azione del Governo c'è stato ed è stato legato alla serietà dell'azione per contenere e combattere la pandemia - che è stata riconosciuta anche dai nostri alleati all'estero, dalle organizzazioni internazionali, dalla comunità scientifica ma non è certo collegato allo stato di emergenza. Peraltro, siamo tutti consapevoli del momento difficile che vivremo in autunno, tutti.

perché in questi mesi sono stati proprio loro a soffrire di più, sradicati da un momento all'altro dai luoghi delle amicizie, dai luoghi dell'apprendimento e della formazione. Davvero su questo abbiamo una responsabilità molto grave,

Il Presidente del Consiglio ha fatto un elenco molto lungo delle cose per cui serve lo stato di emergenza. Ne cito soltanto alcune: strutture temporanee per persone positive, il pagamento delle pensioni delle Poste per gli anziani in sicurezza, la sorveglianza epidemiologica fatta dall'Istituto superiore di sanità, il fatto che il comitato tecnico-scientifico possa continuare il proprio lavoro. Ma davvero, senatore La Russa, pensa che queste siano cose per impaurire gli italiani? Non sono piuttosto cose fatte per rassicurarli? Quindi, senza timidezze e con grande convinzione, il Partito Democratico sosterrà la proroga dello stato di emergenza, per questi motivi, perché serve al Paese, non perché serve a una parte.

spazzare via subito un equivoco che, a mio avviso, sta alla base dell'atteggiamento dell'opposizione. Signor Presidente del Consiglio, lei è un giurista, come ha ricordato anche prima il collega La Russa. Ho ascoltato con attenzione quello che ci ha raccontato la collega Pinotti, quanto sia importante che ci siano dei centri per la cura dei positivi, degli anziani, dei grandi invalidi. Secondo voi, secondo il Governo, tutto questo può essere fatto solamente con il prolungamento dello stato di emergenza? *(Applausi)*. Cioè, secondo voi, l'Italia può essere governata solo attraverso leggi speciali? Questo ci state dicendo?

ci dica poi che questo basta a prolungare lo stato di emergenza per mettere l'Italia sotto leggi eccezionali, dando oltretutto dell'Italia - e qui mi dispiace contraddire i colleghi della maggioranza - un'immagine

Per questo ci opponiamo ferocemente a questa proroga, perché riteniamo che sia, non opportuno, ma doveroso che il Governo si dimostri capace di operare, a prescindere dai pieni poteri che il Presidente del Consiglio e i suoi Ministri vogliono avere grazie allo stato di emergenza. io sono una voce isolata e sono veramente convinta che chi avrà più vantaggio da questo provvedimento sarà lo stesso Governo. La tenuta del Governo La tenuta del Governo sarà politicamente avvantaggiata dal prolungamento dello stato di emergenza ma non l'Italia, gli italiani, l'immagine dell'Italia nel mondo, il famoso *made in Italy* che il ministro Di Maio doveva andare a promuovere in giro per il mondo. *(Applausi)*. Vada a raccontare il ministro Di Maio che promuoviamo un bel prodotto in pieno stato di emergenza. Mi congratulo. Direi che si tratta di un'operazione di *marketing* veramente straordinaria. Anche Anche a livello di consumi interni, signor Presidente, lei ha sentito - lo ha ripetuto oggi l'Istat - che il 30 per cento delle imprese italiane teme di non poter andare avanti. L'unica proroga che lei avrebbe dovuto fare, glielo dico da sei mesi, è la proroga delle scadenze fiscali per i commercianti, gli artigiani e le partite IVA, al 31 di gennaio del 2021. *(Applausi)*. Signor Presidente, non è troppo tardi. È ancora in tempo. Ha fatto pagare una miriade di tasse alle partite IVA a luglio, in questo mese. le chiediamo un ravvedimento operoso ed attivo. Sospenda, proroghi le scadenze fiscali a chi è stato costretto a non lavorare, non ha potuto lavorare perché ha dovuto stare in casa. È solo uno Stato tiranno che chiede di pagare le tasse a chi non ha fatto cassa e deve scegliere se dare da mangiare ai propri figli, pagare i propri dipendenti, i propri fornitori, le utenze, l'affitto o le tasse. Ma è così che si abbassano le saracinesche nelle città. Signor Presidente, io non voglio fare retorica, non voglio raccontare come era il Covid e quanti camion abbiamo visto partire da Bergamo. Tutto questo ci ha colpito terribilmente, ma vogliamo evitare che ricapiti e vogliamo evitare che al resto del mondo l'Italia appaia come un luogo dove tutto questo può ricapitare. Non c'è bisogno dello stato di emergenza per governare bene l'Italia, salvo che non si tratti di un Governo così traballante da avere paura di se stesso, di un Governo che non è in grado di garantire la sanità, la sicurezza, il controllo dell'immigrazione. Ecco: controllo dell'immigrazione, Vogliamo parlare del modo in cui vengono gestite le frontiere Sud, le frontiere del Mediterraneo? Centinaia di immigrati tunisini arrivano in Italia e fuggono dai centri di accoglienza mentre vengono multati i commercianti, gli esercenti che fanno entrare i clienti senza la mascherina. Ci sono immigrati che girano per l'Italia potenzialmente a rischio, perché sappiamo che in Africa, purtroppo, le infrastrutture sanitarie non sono così efficienti. visto che si tratta di immigrazione perlopiù tunisina, una Tunisia che sembra quasi l'Albania degli anni Novanta, io esigo da un Governo come il suo e non significa operare in stato di emergenza, è doveroso - che il Ministro degli esteri richiami l'ambasciatore tunisino per far cessare questi flussi migratori ovviamente mirati ad ottenere qualcosa e si riprenda gli immigrati tunisini che, a parte la rivoluzione dei Gelsomini, non mi risulta siano coinvolti in una guerra. Si tratta di un Paese democratico, civile, che rispetta le convenzioni internazionali, perché dobbiamo tenere centinaia di tunisini a rischio Covid in giro per il nostro Paese? Non abbiamo bisogno del prolungamento dello stato di emergenza per fare questo e comunque temo, visto che non è riuscito a farlo prima, che anche se le prolungheremo lo stato di emergenza, anzi, ve lo prolungherete da soli, sarà difficile farlo anche dopo. Vogliamo parlare delle frontiere del Friuli-Venezia Giulia e la riapertura della rotta balcanica, delle frontiere di Ventimiglia? Sono queste le vere emergenze, signor Presidente del Consiglio, ma non occorre, lo ripeto, invocare diritti e leggi eccezionali per farlo. di norma di grado primario. Allora, per citare e accodarmi a una terminologia giuridica, esiste una norma, la cosiddetta *grundnorm*, la più grande e la più importante di tutte che si chiama Costituzione che dice che il Governo non può limitare per sempre i diritti e le libertà dei cittadini, soprattutto le libertà personali e di esercizio di un'attività economica a rischio ancora adesso. Colleghi, io non so se ci rendiamo conto di quello che stiamo facendo. Qualcuno prima di me - credo il collega Faraone ha invocato lo *smart working*. Ma voi sapete che uno *smart working* che non ha nulla di *smart* sta contribuendo a desertificare le città? Sta contribuendo a impoverire bar e ristoranti non sta assolutamente aumentando la produttività? E noi vogliamo che il nostro Paese rischi che il lavoro si sviluppi in questo modo? Vogliamo far correre alle famiglie e ai lavoratori il rischio di non incentivare il lavoro, che -lo ripeto - è l'unico antidoto alla povertà? Signor Presidente del Consiglio, noi non stiamo creando antidoti alla povertà: un terzo delle famiglie italiane ha risparmi solo per un mese; dall'incrocio dei dati Istat e INPS risulta che negli ultimi due mesi sono state pagate più pensioni che stipendi e questo significa non solo che il *welfare* familiare sta sulle spalle dei nonni, non solo che siamo un popolo di pensionati, ma che, se continua così e se non si incentiva il lavoro, se non si incentivano i salari, tra un po' non pagheremo più neanche le pensioni ai nonni *(Applausi)*. Come facciamo a spiegare a chi ci guarda da fuori e a noi stessi che non stiamo correndo rischi? dopo che avrete dichiarato lo stato di emergenza (è una cosa assolutamente normale che il Presidente del Consiglio venga qui a dirci che dobbiamo essere governati da leggi speciali, altrimenti lei non ne risponde ed è tutta colpa nostra se succede qualcosa), se qualcuno voleva comprare una casa o anche solo una macchina, investire qualche risparmio, anche solo iscriversi e fare un abbonamento da qualche parte, lo farà

che noi non sappiamo, perché non può presentarsi qua dicendo che sostanzialmente i *cluster* Covid sono sotto controllo, che l'incidenza è modesta, ma che lei ha bisogno di governare l'Italia con leggi speciali. Non esiste! Non è possibile fare una dichiarazione del genere, che afferma una cosa e il suo contrario. C'è del metodo nella follia. Lei non riesce a controllare l'immigrazione. Oggi ho visto un'immagine surreale di tunisini che arrivavano con il barboncino

Noi abbiamo paura che tutto questo faccia un danno vero e profondo al lavoro, all'impresa, alle categorie produttive e non siamo soli, parli con il presidente di Confindustria. Lo stato di emergenza non fa bene all'Italia. Chi sa governare governa lo stesso, non ha bisogno di prendersi i pieni poteri, quei pieni poteri che lei contestava l'anno scorso, forse perché era già in predicato di chiederli per sé stesso. Le cito Le cito una frase di qualcuno che sicuramente le piacerà molto, John Kennedy: chi ha cercato di ottenere il potere cavalcando la tigre alla fine viene divorato. Noi Noi stiamo qui, Forza Italia è qui per evitare, per impedire che la tigre dell'emergenza che lei ha scatenato divori il cuore delle categorie produttive, il cuore pulsante, operoso, sano del nostro grande Paese e continueremo sempre ad operare in questa direzione, anche contro di lei

Signor Presidente, ringrazio anche per il mugugno preventivo che mi onora. Si può prorogare lo stato di emergenza? La risposta è negativa e lo è per un motivo molto chiaro, che la situazione di fatto non esiste. Se non c'è uno stato di emergenza, non si può dichiarare l'esistenza di uno stato di emergenza; è stato però obiettato che senza lo stato di emergenza senza emergenza non si possono comprare le mascherine e i banchi per le scuole. Questo argomento, se non fosse comico, sarebbe tragico, perché vorrebbe dire che lo Stato italiano, se non dichiara l'emergenza in assenza di emergenza, non può fare neanche una cosa così semplice come comprare dei banchi monoposto e delle mascherine per gli studenti. *(Applausi)*. Conclusione: la dichiarazione di uno stato di emergenza in questa situazione è inopportuna e illegittima e, quindi, è bene tornare ad una ordinata normalità. Firmato dal professor Sabino Cassese, giudice emerito della Corte costituzionale, che penso che di diritto ne sappia più di lei, professor Conte. Non penso che sia un sovranista o un negazionista perfino banale. Se ci pensiamo, lei ha impiegato quaranta minuti a cercare di dimostrare quello che è indimostrabile e che il professor Cassese smonta in una riga. La dichiarazione è inopportuna illegittima. Ed è grave farsi bocciare all'esame di diritto costituzionale dal professor Cassese con una motivazione semplicissima: senza emergenza non c'è lo stato di emergenza. *(Applausi)*. Lei sta mentendo all'Italia e agli italiani. Lei sta dicendo bugie. Il professor Zangrillo, primario del San Raffaele, ha dichiarato: «Il 18 aprile scorso è stata una data importante. Quel giorno è stato l'ultimo in cui, in un grande istituto ospedaliero di Milano come il nostro, abbiamo avuto un malato grave ricoverato in terapia intensiva col Covid-19. Da allora in poi, non abbiamo più avuto malati con quel tipo di sintomatologia. Da noi, il virus clinicamente non esiste più». Ancora cito il professor Bassetti, direttore della Clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova.

vada a farsi un giro negli ospedali italiani». Cari parlamentari che volete dimostrare il contrario, andate al San Martino di Genova e fatevi accompagnare dal professor Bassetti. L'emergenza c'è solo nella vostra testa ed è un danno per l'Italia e per gli italiani, confermato da chi l'emergenza l'ha combattuta. Non cito il professor Clementi e il professor De Donno, ma cito alcuni colleghi giornalisti, non tutti, ma alcuni, che ogni giorno ci danno il bollettino di guerra. Dedico loro un pensiero di Mark Twain, Mark Twain, che scriveva: il giornalista è colui che distingue il vero dal falso e poi pubblica il falso. In questo periodo storico stiamo assolutamente vivendo in questa verità orwelliana. Questo è il bollettino di oggi. vi sono 40 ricoverati in terapia intensiva. Ieri, su 48.000 tamponi, 181 casi. Oggi, fortunatamente, i morti si sono ridotti a 11. In una giornata media di quest'anno, i morti erano 1.800; una giornata media come quella di oggi, a fronte degli 11 morti, non di Covid-19, ma con il Covid-19, sono morti 658 italiani per malattie cardiovascolari e 485 italiani per tumore. Questi sono i dati che ci fanno ritenere che, se siete gli unici in tutta Europa a prorogare lo stato di emergenza, o non hanno capito niente tutti gli altri o siete in malafede voi. A occhio, siete in malafede voi, perché i numeri questo porterebbero a ritenere. le emergenze vere, a parte il fatto che, sicuramente non un leghista, non un sindaco di centrodestra, ma il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, ha dichiarato ieri: se non lo dichiara il Governo, lo stato di emergenza per Lampedusa lo dichiaro io. E questo stato di emergenza non è legato al Covid-19, ma è legato agli sbarchi che questo Governo, complicemente, sta permettendo, se non organizzando, in questo Paese. Paese. Gli unici turisti che stiamo vedendo, infatti, sono quelli coi cagnolini e i cappellini, che sbarcano a Lampedusa e che poi spariscono per mezza Italia

perché c'è un limite all'incapacità e penso che tale limite sia ampiamente superato. Sono soprattutto le Regioni del Sud che stanno pagando questa vostra complicità: il 17 luglio in 30 scappano da Messina, settimana in 184 scappano da Caltanissetta, in 100 scappano da Porto Empedocle, in 30 scappano da Brindisi, in 23 scappano dall'Umbria, eccetera, eccetera. Temo che ai vertici europei, per farsi regalare qualche prestito, che forse verrà, lei abbia firmato una cambiale in bianco, per tornare a trasformare l'Italia nel campo profughi che l'Italia non si merita. Questi sono i numeri. Se non è forte in diritto costituzionale, lo sia almeno in matematica: 12.000 è più grande di 3.000. A meno che qualcuno non voglia alimentare. Non sono un complottista, però se uno mette in sequenza un comportamento della magistratura vergognoso e indecoroso, perché la giustizia alla Palamara non è la giustizia che si merita il Paese *(Applausi)*, la chiusura delle caserme dei carabinieri, il divieto di manifestare, la proroga dello stato di emergenza, qualche altra sospensione democratica e - perché no? - anche qualche altro rinvio elettorale e magari anche della scelta delle Presidenze delle Commissioni parlamentari, temo che l'unico stato di emergenza che il Paese sta vivendo sia quello della maggioranza di Governo, che non sa più dove sbattere la testa, perché gli italiani vogliono tornare a vivere tranquilli *(Applausi)*. il sovversivo assessore alla pubblica istruzione della Regione Toscana, che temo non sia né salviniano, né leghista, né sovranista, a nome di tutti gli assessori alla scuola, di tutte le Regioni italiane, ha scritto oggi al ministro Azzolina, preoccupato, perché non si sa se, come, quando, con quali fondi, in quali classi e con quali orari riapriranno le scuole italiane. Una delle poche cose che abbiamo capito è che c'è un bando per l'acquisto dei banchi con le rotelle. A proposito di emergenza, l'ABC delle zone sismiche italiane ci insegna che, in caso di terremoto, i bimbi si rifugiano sotto i banchi. Dove si rifugiano i bimbi, se comprate i banchi con le rotelle? *(Applausi)*. E se, Dio non voglia, accade qualcosa, cosa fanno? Il ministro Azzolina non viene attaccato perché è donna e dei 5 Stelle. Il ministro Azzolina viene attaccato perché non è capace di fare il suo lavoro

Mi spiace, perché con la scuola non si scherza! Capisco l'imbarazzo di difendere chi è al posto sbagliato, nel momento sbagliato. L'emergenza, signor Presidente, è quella economica. Domani saranno in piazza i consulenti del lavoro, penso siano una delle categorie più pacifiche, più tranquille, più laboriose e più silenziose della storia italiana, che si sono rotti le scatole di inseguire decreti del Governo, che sono ininterpretabili anche dai professionisti *(Applausi)*. L'emergenza non è legata al Covid-19, ma è legata alla cassa integrazione, che a tanti ancora non è arrivata. Oggi c'erano in piazza i commercianti ambulanti, la settimana scorsa hanno preannunciato lo sciopero fiscale altri pericolosi sovversivi, i dottori commercialisti. Hanno ragione i colleghi del centrodestra: invece di chiudere in casa gli italiani, chiudete nel cassetto i 12 milioni di cartelle esattoriali di Equitalia, che rischiano di essere la mazzata finale per famiglie e imprese. *(Applausi)*. Saldo e stralcio, pace fiscale. Questa è l'emergenza vera: 12 milioni di cartelle esattoriali. L'emergenza sociale denuncia un aumento dell'utilizzo di psicofarmaci e sicuramente chi festeggia in questo periodo sono le grandi case farmaceutiche, a cui magari qualcuno è legato. Non va bene la cura al plasma, perché è democratica e gratuita, ma vanno bene i *business* miliardari delle grandi case farmaceutiche. Amici dei 5 Stelle, siete finiti male. *(Applausi)*. Dalla Dalla difesa del popolo sovrano, alla difesa dell'interesse delle multinazionali del farmaco: che triste fine. Ma ognuno raccoglie quello che semina. Sul turismo... Tempo? Penso di aver diritto di concludere il discorso, se non è troppo. eccezionali questa maggioranza e questo Governo, che non solo vogliono imporre una verità che non esiste, ma pretendono anche che tutto il popolo italiano plauda gaudente la loro verità che non esiste. *(Applausi)*. Noi rappresentiamo l'Italia delle donne e degli uomini liberi. Se vi dà fastidio, uscite da quest'Aula, visto che siamo comunque maggioranza nel Paese e torneremo a essere maggioranza anche in quest'Assemblea del Parlamento. *(Applausi)*. Perché prima o poi gli italiani voteranno, senza mascherina e dandosi la mano.

Ognuno raccoglie quello che semina. Se voi pensate di imbavagliare gli italiani, con la strategia della paura e della chiusura, sbagliate, perché fate il male del Paese. L'immagine che mi piace di questo Paese è quella di Beatrice Vittoria, che è nata due giorni fa all'ospedale di Mantova da una mamma che è guarita dal Covid-19, grazie alla cura al plasma del dottor De Donno, e rappresenta quelle italiane e quegli italiani che non si arrendono e che non fanno finta di credere alle menzogne che voi cercate di propinarci a reti unificate. *(Applausi)*. Viva l'Italia, viva la libertà, viva la gente che ha voglia di amare e lavorare tranquillamente.

da tutte le parti.

lo stato d'emergenza; ci ha illuminato sul problema di carattere tecnico che riveste la proroga, sul fatto che si tratta solamente di un potere di ordinanza della Protezione civile in base al decreto legislativo n.

Ci sono anche altri casi di stato d'emergenza che potremmo citare: per esempio, nel 2003, con il secondo Governo Berlusconi, fu dichiarato lo stato di emergenza nazionale per il delicato panorama internazionale conseguente alla guerra in Iraq. Mi sembra che all'epoca ci fossero come ministri sia il senatore Gasparri che il senatore Calderoli, quindi forse un po' se ne intendono e possono illuminare il centrodestra su cosa significhi lo stato di emergenza. Ancora, nel 2010 fu dichiarato lo stato di emergenza per la SARS, e mi sembra che anche in quel caso fosse ministro il senatore La Russa. È molto singolare, poi, sentir dire,

lui. È così interessante sentir parlare del tema della paura. Il presidente Conte ci ha ricordato che non vogliamo assolutamente alimentare la paura, tema giusto e sacrosanto, perché non è con la paura che si fanno le cose. A tal proposito voglio leggere un passaggio interessante che cita queste parole: «Eravamo già ciechi nel momento in cui lo siamo diventati, la paura ci ha accecato, la paura ci manterrà ciechi». Si tratta di un

giorno. Forse questo ci fa capire che un virus di questo tipo interviene a livello globale, e se c'è stato il picco dei contagi in un solo giorno potrebbe esserci un problema di ritorno del virus. A questo punto dobbiamo ringraziare non solo il Governo, ma soprattutto i cittadini italiani, che sono stati molto attenti utilizzando le mascherine per fare in modo che il contagio non si diffondesse. *(Applausi)*. Questo è veramente un merito che dobbiamo attribuire ai nostri cittadini.

Ed è al livello globale che ci dobbiamo confrontare perché dobbiamo capire che il virus viaggia velocemente e quanto è importante stare attenti a tutto ciò che facciamo. Il virus ci ha messo di fronte a un bivio importante. Nel mondo c'è stato un momento in cui si è verificato un cambio di direzione. Era la fine della Seconda guerra mondiale; c'è stata la Prima guerra mondiale, poi c'è stata la crisi del 1929, la Seconda guerra mondiale e, in quel momento storico, c'è stato un cambio di direzione. Noi dobbiamo ricordare la storia perché grazie ad essa riusciamo a capire realmente qual è la strada che abbiamo davanti. Abbiamo davanti una strada in cui il neoliberismo che ha dominato il sistema politico internazionale, in cui sono aumentate incredibilmente le disuguaglianze, quel neoliberismo che è giunto ad un momento di crisi, ha prodotto anche delle conseguenze molto particolari. Basterebbe citare qualche dato. Un elemento interessante lo possiamo trarre leggendo i valori di capitalizzazione di alcune aziende. Vi faccio qualche esempio. Apple capitalizza 1.636 miliardi di dollari, Microsoft 1.500, lo stesso Amazon, Alphabet 1.044. Queste quattro società da sole capitalizzano 5.754 miliardi di dollari, più del PIL del Giappone, che è il terzo Stato per PIL del mondo e queste società hanno tutte sede in un paradiso fiscale. Allora forse dovremmo capire qual è l'obiettivo e comprendere che c'è bisogno di uno Stato più forte, c'è bisogno che i Governi e i popoli si riprendano la loro sovranità per cercare di dire a queste società che quello che dobbiamo fare è l'interesse collettivo e non quello delle singole società. Oltre tutto queste società hanno tutte sede in un paradiso fiscale; quelle statunitensi hanno sede nel Delaware, quelle cinesi, tra cui, per esempio, Alibaba, ha sede alle Isole Cayman. Questo è un altro tema con il quale ci dobbiamo confrontare; la lotta ai paradisi fiscali, che non sono solo quelli internazionali. Ci sono i paradisi fiscali intracomunitari con i quali dobbiamo combattere e verso i quali dobbiamo rivolgere la nostra attenzione. Nel momento storico di cui parlavo prima

aveva studiato il comportamento degli animali in Siberia e si contrapponeva alle teorie darwiniane, spiegando che, in situazioni di carenza di risorse, solo la cooperazione fra le persone, in quel caso la cooperazione tra animali, rendeva forte la specie.

un sistema diverso poteva cambiare il mondo. Ci troviamo di fronte ancora una volta al fatto che non capiamo, siamo ciechi, come diceva Saramago, di fronte alle realtà che viviamo: quando vediamo che in Antartide si arriva a 20 gradi, forse dovremmo iniziare a capire che questa è la strada da percorrere. Dobbiamo aprire gli occhi, dobbiamo renderci conto della situazione nella quale siamo, perché solo così impostiamo una nuova strategia politica, un nuovo percorso, che è quello che il Governo sta cercando di realizzare con tutte le sue forze e l'intera maggioranza è compatta nel sostenere questa azione, per immaginare un mondo che sia diverso, in cui ci sia una forza che si contrapponga al totale liberismo, che ha dominato negli ultimi quaranta

queste cose, raccontare la storia, però è sempre molto interessante capire qual è la realtà. Ci troviamo di fronte a questa realtà e questa è la strada che noi vogliamo intraprendere, questa è l'azione politica che noi vogliamo mettere in campo perché in questa sede dobbiamo parlare anche di politica. La nostra strada, che tutti quanti auspichiamo, ci porta verso un modo diverso

Non ci può essere libertà senza giustizia sociale e non ci può essere giustizia sociale senza libertà, perché - altrimenti - è solamente la libertà di morire di fame. Queste sono le parole che sono al centro dell'azione del Governo e della maggioranza: equità e giustizia sociale, associate al tema delle libertà. *(Applausi)*. Questa è la direzione verso la quale stiamo andando e questo è il supporto dell'intera maggioranza nei confronti del Governo. E se c'è bisogno dello stato di proroga, noi siamo completamente convinti che sia utile e necessario.

non sono tra coloro che sostengono che la proroga dello stato di emergenza sottenda a delle pressioni antidemocratiche autoritarie, né tantomeno tra chi - canagliescamente - ha sostenuto che il Governo sparga infetti per giustificare i provvedimenti antidemocratici. Tuttavia, è un fatto che la proroga di cui stiamo discutendo porterà con sé anche la proroga di strumenti straordinari, come ordinanze e decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Questa situazione, se era accettabile nel momento in cui la pandemia aveva tutta la sua forza e virulenza, oggi - a mio giudizio - non lo è più. A chi ricorda che ci sono stati molti altri stati di emergenza, ricordo che - però - questa è la prima volta che il Parlamento delega il Governo a disciplinare con meri atti amministrativi i diritti fondamentali dei cittadini. Ripeto che questo poteva essere tollerabile nel picco della pandemia, mentre oggi non lo è più. Con ciò non intendo che si debba abbassare la guardia, ma ritornare nell'alveo della Costituzione e disciplinare ciò che è necessario con gli strumenti ordinari, anche d'urgenza, come ad esempio i decreti-legge. Dico questo perché temo che la maggioranza stia consegnando ai posteri un precedente pericoloso,

ha subappaltato la gestione dell'emergenza a tecnici o presunti tali, che non sono mai stati scelti dai cittadini per affrontare le sfide della nostra Nazione. Il dato tuttavia più grave di questa vicenda è l'assoluta incapacità del Governo nella gestione di questa emergenza. È stato più volte detto che non torneremo alla normalità, perché non c'è una cura, e che torneremo alla normalità solo quando avremo un vaccino. Ebbene, una cura è stata già citata, quella del plasma iperimmune del professor De Donno; è fantastico che poi siano stati donati dal presidente Conte e dal Governo milioni di euro alla Gavi Foundation di *mister* Bill Gates, mentre invece al professor De Donno sono stati inviati i NAS. Questi sono i fatti.

Mi hanno riso dietro e alcuni mi hanno dato ragione, perché avevo chiesto di sperimentare e di valutare l'opportunità dell'utilizzo della cannabis medica. Ebbene, qualche giornale mi ha riso dietro.

metabolita non psicoattivo della Cannabis sativa,» - quindi può piacere a voi - «può aiutare a ridurre la tempesta citochimica e l'eccessiva infiammazione polmonare che si è rivelata letale per molti pazienti con Covid-19. (...) potrebbe aiutare i pazienti con difficoltà respiratorie evitando trattamenti come la ventilazione meccanica e riducendo i rischi di morte». In Olanda, signor Presidente, dall'inizio del *lockdown*, se non hai sintomi per ventiquattro ore sei guarito; in Italia teniamo in casa i debolmente positivi. C'è una bambina dell'*hinterland* milanese che è a casa da quattro mesi, perché risulta essere debolmente positiva e i tamponi sono tutti contraddittori. Una volta è positiva e una volta è negativa; non esce di casa perché secondo voi e secondo la *task force* ce ne vogliono due consecutivi negativi. Oggi, con questa proroga con questi provvedimenti, senza alcuna visione del futuro, distruggiamo le casse pubbliche per avvantaggiare i soliti noti. Concludo: stiamo ipotecando il futuro dei nostri ragazzi. Per questi motivi voterò contro la proposta di risoluzione della maggioranza.

Perché questa emergenza, numeri alla mano, esiste solo nelle vostre teste. Chiamate malati da mettere in quarantena persone sane e asintomatiche, per le quali i tamponi fatti successivamente hanno dato esiti contraddittori.

Fate migliaia di tamponi ogni giorno, pur di poter alzare il numero dei contagiati; e parlate di contagiati come se fossero malati. I contagiati non sono malati. *(Applausi)*. che l'etica professionale insegna che non si deve trasformare in malato una persona che non lo è. Ippocrate diceva questo e i medici fanno un giuramento su questo. È stato citato il caso dell'Olanda, dove, dopo ventiquattro ore di non sintomaticità, sei guarito e non contagioso. Allora, o il virus olandese è come Lupo de' Lupis, il virus tanto buonino, oppure gli olandesi sono fessi oppure c'è qualcosa che non va. Per finire, avete imposto protocolli che classificano come morto Covid praticamente chiunque. Nonostante questo, il numero dei morti giornalieri è inferiore al numero dei suicidi in Italia. Questa è l'emergenza. Avete coniato, grazie alla stampa, il termine negazionista, per etichettare, quando non avete argomenti, persone che hanno un pensiero proprio argomentato. Per esempio, Zangrillo improvvisamente è diventato un negazionista, cioè una persona da mettere a tacere. Questa non è democrazia. Citando uno psicologo, questo è fascismo sanitario, per cui bisogna dire basta: gli italiani devono tornare a vivere e liberarsi dal cappio che continuate a tenere loro sulla testa. Basta!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

n. 2, presentata dai senatori Romeo, Bernini e Ciriani, col parere contrario del Governo, risultano preclusi tutta la prima parte (le premesse) e il primo capoverso «a non procedere alla proroga dello stato di emergenza», eccetera. Rimane assorbito il secondo capoverso, da «qualora l'andamento della situazione epidemiologica»

un procedimento normativo che prevede anche che siano sentiti «i Presidenti delle Regioni interessate, nel caso in cui le misure riguardino esclusivamente una Regione o alcune specifiche Regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale», propongo di mettere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

un evento storico importante che quarant'anni fa si è celebrato e ha visto un italiano, un mio concittadino di Barletta, salire sul tetto del mondo.

Signor Presidente, colleghe e colleghi, negli ultimi tempi la provincia in cui vivo, Belluno, è colpita duramente da un numero elevato di predazioni del lupo, tant'è che è ormai diventata cronaca quotidiana. La situazione non è diversa nell'altopiano di Asiago, sulla Lessinia e nelle province limitrofe. La settimana scorsa ho ricevuto molte telefonate da allevatori che mi hanno manifestato il loro sconforto per quanto sta accadendo ai loro capi di bestiame, sbranati o feriti a morte.

Ero talmente incredulo che sono andato a trovare uno di questi allevatori e purtroppo la conferma è stata netta. Credo sia davvero inaccettabile che questa situazione, che dovrebbe essere gestita con accuratezza per garantire un sano equilibrio tra ambiente e uomo, passi nella totale indifferenza dei rappresentanti di questo Governo.

a incontrare le persone coinvolte per comprendere la gravità della situazione. C'è un aspetto economico da considerare, che è quello del rischio della scomparsa dell'intera filiera agroalimentare del territorio, al quale si aggiunge la possibile chiusura delle attività da parte degli allevatori. Ma non meno importante è l'aspetto della sicurezza del cittadino. I cani e i gatti sono animali domestici che in linea di massima stanno nel cortile o nel giardino di casa, e non all'interno di un recinto, giocando magari con bambini e persone. Altrettanto serio è l'aspetto dell'affettività uomo-animale: proprio l'altro giorno ho visto gli occhi pieni di lacrime di una bimba che accarezzava la sua piccola pecora agonizzante dalle ferite; animale del quale si era presa cura lei stessa. Voglio concludere con una considerazione di una cittadina dell'Alpago, terra da cui provengo, che dice: «Bisogna aiutare gli allevatori a risolvere questo problema, vorrei che tornasse l'armonia e la tranquillità di un tempo». Se i lupi sono stati messi per predare i cervi, mi sembra che il progetto stia fallendo. Non aspettiamo che ci sia l'estinzione della pecora alpagota, razza autoctona locale e...

Signor Presidente, mi sia consentito un breve ricordo di Gianrico Tedeschi, un attore molto amato, la cui scomparsa, avvenuta ieri all'età di cento anni, è una perdita per il mondo della cultura e per tutto l'antifascismo italiano. Quando, nel novembre dello scorso anno, il professor Luciano Zani mi propose di raccogliere la storia dell'attore nel ciclo di incontri che la biblioteca del Senato aveva voluto dedicare alle vicende degli internati militari italiani, mi parve un tributo meritato e necessario. Tedeschi, che oggi commemoriamo all'indomani della sua scomparsa, fu uno degli 800.000 soldati catturati dalla Wehrmacht dopo l'8 settembre del 1943. Partì per il fronte greco nel 1941, quando aveva ventuno anni ed era uno studente di lettere, un sottotenente intelligente e simpatico. Arrestato nell'autunno del 1943 non aderì alla Repubblica sociale italiana e scelse di affrontare la prigionia. I libri che nel novembre scorso presentammo nel Palazzo della Minerva hanno il merito di ricostruire i due anni di prigionia scontati dall'attore in diversi *lager* tra i quali Sandbostel e di come l'amore per il teatro lo abbia aiutato nella difficile impresa della sopravvivenza. Più volte gli internati militari italiani hanno infatti ricordato come nei campi di internamento la salute spirituale fosse importante quanto quella del corpo. Tedeschi, come altri protagonisti di quel periodo - su tutti ricordo il partigiano "Geppe", Nino Garau, anch'esso recentemente scomparso - scelse di non rendere subito nota quell'esperienza: un percorso difficile e doloroso quello dell'internato, che l'attore ebbe bisogno di elaborare, sminuzzare, digerire prima di poterlo condividere. Condivise, alla fine, questa esperienza dei *lager* con altri intellettuali del calibro di Giovannino Guareschi, Alessandro Natta, Giuseppe Lazzati, Arturo Coppola, Giuseppe Novello, Roberto Rebora ed Enzo Pace. Ognuno di essi ne fece esperienza decisiva per l'impegno a favore di un'Italia democratica più giusta e lontana dalle tenebre del pensiero nazifascista. In lui, in Gianrico Tedeschi, a cui va il tributo mio e credo dell'intera Assemblea di Palazzo Madama, restò sempre vivido il disagio per gli anni immediatamente successivi alla Liberazione, quando, per un certo tempo, la scelta coraggiosa, cioè il rifiuto dell'adesione degli internati militari della Repubblica sociale, non venne adeguatamente valorizzato. Molti di loro patirono un'ingiusta discriminazione, oggi finalmente superata.

Cara presidente Alberti Casellati, il suo richiamo è stato più che legittimo. Tuttavia, avrebbe potuto farlo alla fine, ma evidentemente per lei, cara Presidente, è stato talmente necessario, questo richiamo, da scippare per un paio di minuti la scena al nostro Presidente del Consiglio durante un'informativa di una giornata, per l'Italia, destinata a restare nella storia. Mi accordi, tuttavia, di dirle che il suo richiamo alle regole è stato più dannoso del fatto in sé, ovvero dell'aver immortalato con lo *smartphone* e non con la macchina fotografica quel momento storico. Dannoso ed aggiungo irriverente, nei confronti del presidente Conte e di tutti quegli italiani che seguivano la diretta televisiva Rai. Concludo esortandola alla coerenza: che futuri richiami siano fatti in modo nominale, proprio come ha fatto con me e con la collega Botto, soprattutto per non risultare scortese nei confronti di tutti quegli altri colleghi che, come me, in quella circostanza hanno fatto foto e video, magari di altri schieramenti che oggi sono pure all'opposizione e che fino ad ora non hanno mai avuto lo stesso privilegio di essere richiamati nominalmente durante una diretta televisiva, provocando l'interruzione di un'informativa del Presidente del Consiglio. Le regole sono regole, ma valgono per tutti. Vorrei ricordarle semplicemente che io ho aspettato, come lei ricorderà perfettamente, che il Presidente del Consiglio

quando doveva ricominciare a parlare e c'era una senatrice, un'altra sua collega che lo aveva fatto precedentemente e continuava a fare delle foto. Io ho aspettato questo momento proprio per non interrompere il Presidente del Consiglio. Dall'altra parte, però, le vorrei ricordare che forse, siccome c'è un Regolamento che parla chiaro e che tutti voi senatori dovreste conoscere, non dovrei neppure essere in nessuna occasione, che ci sia una diretta televisiva, nella necessità di richiamare all'ordine sul Regolamento che dovrebbe essere da tutti conosciuto. Pertanto io mi sarei risparmiata volentieri questo, se non ci fosse stato un atteggiamento ripetuto, perché non avevo interrotto; la sua collega era lì, in mezzo all'Emiciclo, continuava a fotografare, era stata segnalata e avevo lasciato stare, poi ha cominciato lei e pertanto, quando è finito l'applauso, vi ho richiamato come va fatto. Infatti, va fatto nominalmente, come da voi è sempre richiesto quando lo fanno gli altri, tanto è vero che, come lei ricorderà, avevo sollecitato, quando voi protestavate perché qualcuno faceva fotografie, di dirmi il nome, perché non riuscivo ad individuarlo.

che contravvengono alle regole, perché ho richiamato sempre tutti, da una parte e dall'altra. Pertanto, penso di averle spiegato che non c'era nessuna intenzione di rovinare - lei mi dice - questo momento importante.

Senatore Perilli, trovo inaccettabile questo suo comportamento davvero irrispettoso. Io ho risposto in maniera molto educata alla gentile senatrice,